Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana a seguito della scomparsa del senatore Altero Matteoli, ha riscontrato, nella seduta del 20 dicembre, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Franco Mugnai. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Franco Mugnai. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Signor Presidente, i colleghi sanno che stiamo per approvare la legge sui testimoni di giustizia

di giustizia, ma per i collaboratori di giustizia. Ricordo a tutti i colleghi che si era in una fase storica in cui lo Stato italiano per la prima volta decideva di sfidare le mafie,

che fanno il loro lavoro, che vengono a conoscenza di fatti di mafia e che, piuttosto che girare le spalle, negare e far finta di non vedere, decidono di fare il loro dovere di cittadini, cioè

bestia le mafie, che nei confronti di un cittadino onesto che testimonia non accettano l'idea che qualcuno possa inserirsi in un affare che non gli appartiene, mafie l'omertà è il cardine della relazione con i cittadini onesti: «Fatti i fatti tuoi. Non ti immischiare, non sono questioni che ti riguardano».

cui la mattina danno il loro contributo e già la sera devono abbandonare la loro vita reale e il loro lavoro: allontanarsi dalla propria abitazione, interrompere tutti i rapporti con gli amici, portare i loro figli via dalla scuola

c'è il passaggio successivo di consentire ai testimoni di giustizia di potersi reinserire nella vita reale, perché la testimonianza è un tratto della propria vita, non è la vita: la vita sono il lavoro, le relazioni, la famiglia e il territorio e tutto questo deve essere fatto in condizioni di anonimato, addirittura cambiando le proprie generalità. Immaginate una persona che, tutto ad un tratto, ha un altro nome e un altro cognome e noi sappiamo che l'identità

capire bene la portata di quella decisione e senza comprendere bene perché il loro papà e la loro mamma li hanno portati a fare quella scelta.

vale anche per altri familiari che, il più delle volte, diventano oggetto di ritorsione e di vendetta, per cui è su costoro, che rimangono nella località di origine, che si scatenano la furia e la violenza mafiosa abbiamo avuto molti casi che ci mostrano che quella scelta è stata sottoposta poi ad un elevato sacrificio).

che parte sin dall'origine dall'idea che il testimone di giustizia è una risorsa e non un problema per lo Stato italiano ed è una risorsa preziosa. Per questo dobbiamo chiedere scusa ai testimoni di giustizia. Dobbiamo capire che abbiamo fatto degli errori gravi e che adesso possiamo finalmente compiere una scelta che ci consenta di guardarli negli occhi, come Stato che dà la mano al proprio cittadino ed insieme ad essi compie delle scelte serie, in grado di portare a degli impegni che possano essere mantenuti.

d'origine. Questa è un'altra scelta dirompente, di rottura. Lo Stato, come prima opzione, deve consentire a chi fa il testimone di giustizia di non essere sradicato. Naturalmente va valutato il pericolo reale e, in proporzione al pericolo reale, lo Stato deve fare di tutto perché il testimone sia tutelato e la sua attività economica, sociale, affettiva e familiare possa esplicarsi lì egli ha vissuto, dove ha maturato questa scelta e dove deve diventare un esempio per tutta la comunità locale e per gli altri cittadini. Oggi anche questa opzione che, normativamente, prima era secondaria - anzi era quasi bistrattata - diventa una opzione alla pari di quella che si consuma quando il testimone viene portato via dalla propria località. Quindi, gli articoli scorrono lungo questo filo: il testimone come risorsa, risorsa rimanendo nel luogo di origine, risorsa quando è costretto, per motivi di protezione, ad essere allontanato, risorsa, non solo quando testimonia, ma anche quando deve essere reinserito nella vita sociale; anche quando deve essere protetto con delle norme di sicurezza che non sono a fisarmonica: di grande rilievo quando si testimonia e poi, alla fine, sempre più ridotte, addirittura poi venendo meno quando si finisce di dare questa testimonianza. Abbiamo avuto dei casi gravissimi. Pensate al caso Lea Garofalo, casi in cui poi le mafie, che non dimenticano, sono intervenute e hanno causato lutti e dolori immani a quelle persone e ai loro familiari. Anche questo viene superato perché il sistema di sicurezza deve essere sempre allerta, proporzionato, vigile e non deve essere strumentale per usare testimoni e poi abbandonarli al loro destino. Con queste scelte, cari colleghi, possiamo arricchire la legislazione antimafia di questo altro strumento. Signor Presidente, lei sa che questa è stata una legislatura molto ricca di interventi proprio nel campo della lotta alle mafie. Non era mai successo che finalmente ci si spostasse dall'antimafia del giorno dopo (quella emergenziale, quella che rincorre gli atti spesso violenti e le stragi delle mafie) cercando di avanzare verso l'antimafia del giorno prima (quella che anticipa, quella che comprende, quella che finalmente dà allo Stato la possibilità di dettare i tempi). Certo, siamo ancora all'inizio dell'antimafia del giorno prima. Ancora c'è bisogno di ulteriori interventi e c'è bisogno ancora di migliorare il nostro sistema sia culturale sia giuridico, che operativo, ma è la strada che abbiamo imboccato in questa legislatura e ha bisogno, quindi, di andare avanti, di esplicare tutte le proprie potenzialità. Vi assicuro, però,

ritengo che l'aspetto giuridico sia ovviamente importante, perché non si può discutere di un testo legislativo senza valorizzarne gli aspetti in diritto, però ritengo che l'aspetto politico sia addirittura preminente. Parliamo dei due versanti sui quali occorre intrattenersi. Intanto vi è un versante soggettivo, ossia di individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli dei criteri del sistema di protezione, delle tutele introdotte da questa legge. Da questo punto di vista c'è una dilatazione importante, perché non si comprendono soltanto i testimoni di giustizia, ossia coloro i quali hanno svolto

responsabile alla qualità delle dichiarazioni, perché c'era un problema costituito dalla necessità di individualizzare il trattamento riservato ai testimoni di giustizia a coloro i quali risultassero meritevoli. Qui l'obiettivo è perseguito su di un doppio versante. Per un verso, si dice che costoro debbano avere reso delle dichiarazioni attendibili in senso intrinseco, e per giunta fondatamente attendibili. C'è l'utilizzazione di un attributo che forse poteva ritenersi superfluo, quella della fondatezza dell'attendibilità, perché si sarebbe potuto obiettare che ciò che è attendibile lo è in quanto è fondatamente attendibile. Però l'uso, forse enfatico, plurimo, dell'attribuzione serve a sottolineare che non si può pretendere di beneficiare di un trattamento di questo genere solo per aver reso delle dichiarazioni che magari si collocano in un'area di dubbio. Quindi parliamo di attendibilità per giunta oggettiva, perché l'altro attributo, quello dell'attendibilità intrinseca, è derivato da una collaudata dal 1991, perlomeno con la prima sentenza a sezioni unite, quella relativa all'omicidio del commissario Calabresi) secondo la connotazione intrinseca oggettiva della dichiarazione. Quindi essa viene dopo l'attendibilità soggettiva e costituisce un corredo rassicurante della circostanza che quel soggetto merita effettivamente la protezione che gli viene riservata. lo diceva il relatore, vi è un aspetto di umanizzazione della tutela, perché la tutela non può spingersi, salvo il caso in cui vi siano delle prevalenti esigenze di sicurezza, fino al punto di allontanare questi soggetti dal luogo in cui essi vivono e dove esercitano quelle attività lavorative che costituiscono il loro sostegno e della loro stessa famiglia. linea principale, vi è il diritto a rimanere nel posto dove si vive, dove si intrattengono le proprie relazioni lavorative, sociali e umane, salvo che non siano prevalenti quelle esigenze di sicurezza che eventualmente possano possano consigliare l'allontanamento da quei posti; e poi il diritto al mantenimento delle relazioni affettive che costituisce un necessario *pendant* rispetto al diritto a rimanere là dove si è sempre vissuti. Dicevo, l'altro parametro a mezzo del quale si persegue l'obiettivo di garantire dichiarazioni attendibili è costituito dalla introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, a corredo del delitto di calunnia, per coloro i quali abbiano, nel tentativo di ottenere ovvero di permanere sotto il regime di speciale protezione, reso dichiarazioni false nella consapevolezza della loro falsità, quindi attribuendo un fatto ad un soggetto il quale si sapeva prima ancora essere innocente. Le misure ulteriori sono volte un sostegno economico che, avvedutamente, centra l'obiettivo del mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello al quale è si è rinunciato. Dicevo in apertura (e sarei incompleto se non dessi conto di quest'altro versante) che la scelta politica è in un certo senso sovrastante dal punto di vista valoriale e di quelle ragioni che dirigono la decisione del legislatore in una direzione o in un'altra rispetto al pur cospicuo e altrettanto rilevante versante giuridico, ossia in cosa le scelte assiologiche del legislatore si sono poi concretizzate. discussione interveniamo infatti su quello che potrei definire lo snodo essenziale di ogni buona democrazia, ossia i fatti regolativi del rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Questo è uno degli elementi fondamentali della democrazia, perché il cittadino rinuncia a determinate sue prerogative, anche di libertà, nei confronti di uno Stato il quale assolva

Lo Stato si assume quindi obblighi di tutela nei confronti dei cittadini, consistenti nell'assicurare le migliori condizioni di vita, e si obbliga a mantenere la pace e la coesione sociale, in cambio di una cessione di diritti individuali del cittadino. Non era quindi pensabile che, in un contesto che costituisce l'in sé del rapporto di fiducia e quindi delle garanzie democratiche, lo Stato venisse meno ad un obbligo di solidarietà nei confronti di soggetti che rinunciano alla loro tranquillità familiare, al diritto di vivere laddove sono nati, ai rapporti affettivi, sociali, ai vantaggi economici conseguenti a un'attività che loro hanno liberamente esercitato da sempre. Non era ipotizzabile uno Stato renitente, omissivo e latitante nell'assolvere ai suoi doveri, non soltanto di protezione ma anche di garanzia, in ordine alla prosecuzione e al mantenimento di condizioni di vita l'assunzione di un obbligo importante da parte del cittadino nei confronti dello Stato, che si sostanzia nell'obbligo di rendere leale il proprio comportamento nei confronti dello Stato stesso e nell'assolvimento di un difficile ma doveroso obbligo di lealtà nei confronti dell'amministrazione della giustizia, rendendosi protagonisti di un comportamento assolutamente fedele ed osservante rispetto alle regole, con ciò assumendosi rischi non soltanto

regolativi di questo difficile rapporto tra Stato e cittadini, che questo testo normativo realizza in un contesto di realtà e di assolvimento reciproco di obblighi. In questa direzione credo che il testo meriti

quella esibizione inutile di chi dice le stesse cose in discussione generale e in dichiarazione di voto di anticipare in questo sia pur differenziato contesto il voto favorevole del Gruppo al quale sono iscritto.

che ha sostanzialmente esteso ai testimoni di giustizia le misure a favore dei cosiddetti pentiti e qualcuno potrebbe pensare che, essendoci già una legge, sia superfluo approvarne un'altra. In questo tempo ci si è resi conto che molte situazioni andavano normate meglio, a partire dalla definizione di testimone che è stata indicata dal decreto-legge n. 8 del 1991 che ha esteso a loro alcuni ambiti di premialità dei collaboratori di giustizia. Basandosi su un'analisi superficiale sembrerebbe che le due figure, avendo alcuni tratti in comune, non necessitino di specifiche e che la normativa fosse più che sufficiente. Invece, analizzando lo stato attuale sono emerse diverse criticità che possiamo riassumere in un massiccio ricorso ai programmi di protezione in località protetta, in situazioni spesso degradate e in completo isolamento sociale, un'insufficienza delle risorse economiche e in una disparità di trattamento tra testimoni di giustizia e, infine, in un'eccessiva rigidità delle procedure. Proprio per superare queste criticità che è stato predisposto e approvato alla Camera questo provvedimento, che oggi ci accingiamo a licenziare. Tra i punti salienti di questo disegno di legge segnalo il riconoscimento della protezione delle persone conviventi ai testimoni e una migliore definizione giuridica. Si definiscono le tipologie delle speciali misure di protezione, che si sostanziano in misure di tutela fisica, economica e di inserimento sociale e lavorativo. Si precisa che le misure di protezione dovranno essere personalizzate, indipendentemente se adottate nella località di origine o in quella protetta. Anche il sostegno economico viene articolato per andare incontro alle necessità del testimone e dei suoi familiari: gli viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, come il diritto ad un alloggio di pari dignità, il diritto a un'assistenza legale e un indennizzo forfetario; nel caso di trasferimento in un luogo protetto, lo Stato acquisterà poi i suoi immobili, corrispondendo il denaro ai testimoni. Altro aspetto innovativo consiste nell'individuazione delle misure di reinserimento sociale lavorativo, che prevedono la possibilità di accesso a un'attività lavorativa anche non retribuita, la possibilità di beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa e la possibilità di accesso alla gestione di beni confiscati. Questa legge, oltre a tutelare gli interessi economici e sociali del testimone, si concentra anche sul versante istituzionale, innovando la composizione della commissione centrale, e del Servizio centrale di protezione, merito alle proposte di ammissione alle specifiche misure di protezione. Si semplifica inoltre la disciplina del piano provvisorio e definitivo di protezione. Importante e forse la novità maggiore di questo provvedimento è l'articolo 16 che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale. Va specificato che il referente ha compito esclusivamente assistenziale e che la titolarità della decisione resta comunque in capo al testimone. un lato mette al centro il bisogno del testimone, tant'è vero che in stato di necessità potrà interloquire direttamente con la commissione centrale; dall'altro lato lo responsabilizza ulteriormente: in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere illeciti benefici scatta un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia. Concludo, Presidente, dicendo che questa sarà una buona legge che sanerà distorsioni del passato e ridarà fiducia a persone che hanno dato molto a tutti noi e che spesso non hanno ricevuto in proporzione. una legge che per me assumerà un significato speciale: sentire con le proprie orecchie le emozioni, l'ansia e la fatica del vivere dei testimoni di giustizia resterà un ricordo indelebile. Spero che sia data grande visibilità al provvedimento, perché la sua conoscenza potrà incoraggiare altri cittadini a denunciare. *(Applausi

con un sistema di garanzie sia sotto il profilo della tutela personale sia sotto il profilo degli aiuti economici sia sotto il profilo del sostegno psicologico e altro quello che interessa di più è che questo disegno di legge finalmente riconosce il ruolo che i testimoni di giustizia hanno nel garantire, con le loro dichiarazioni, un contributo effettivo all'accertamento delle responsabilità. Vi è tutto un sistema di garanzie che vengono attuate e, allo stesso tempo, come è stato appena ricordato dal collega del Movimento 5 Stelle, c'è

questo provvedimento segni un discrimine tra la buona politica e la cattiva politica. La buona politica affronta

vita. Innanzitutto occorre segnare la differenza tra costoro e la figura del collaboratore di giustizia, perché questa sovrapposizione troppo spesso, nel linguaggio comune, rischia di non aiutarci a mettere a fuoco di chi stiamo parlando. Il testimone di giustizia non è il pentito e non è persona che si sia macchiata di qualche crimine e abbia deciso di collaborare. Il testimone di giustizia è persona assolutamente innocente che decide di mettersi a disposizione dello Stato. Quando parliamo del fenomeno dell'omertà in alcune zone del nostro Paese, dobbiamo avere sempre molto chiaro qual è il destino, qual è il contesto in cui si va ad inserire la persona che decide di sfidare il silenzio, che decide di denunciare. Questa persona si mette nelle mani di uno Stato che spesso non è in grado di difenderla. Con questa legge rendiamo più facile difendere la figura del testimone di giustizia a partire da una innovazione importante, una delle più importanti, credo, contenuta all'interno

di trasferimento in luogo protetto, che devono rimanere l'ultima *ratio* considerato l'impatto formidabile che hanno sulla vita di queste persone. Segnalo poi le modificazioni che ci sono anche rispetto alle previsioni: la possibilità di assunzione nella pubblica amministrazione e le possibilità a favore delle

Ancora, è importante la possibilità di utilizzo dell'incidente probatorio e della videoconferenza per ascoltare queste persone, la cui sovraesposizione va assolutamente evitata proprio per il rispetto del pericolo cui stanno esponendo

che sia un atto dovuto, da parte di questo Parlamento, riuscire, in questo finale di legislatura, a portare a termine una promessa, che non è solamente nei confronti di queste persone, e non è solamente nei confronti di quelle organizzazioni della società civile che tanto hanno premuto ma è anche e soprattutto volta ad impegnarsi a realizzare uno dei principi costituzionali più caratterizzanti, cioè il rispetto della legge. Il rispetto della legalità richiede sostegno a chi si faccia carico, mettendo in gioco la propria esperienza, la propria esistenza, la sicurezza della propria famiglia, di aiutare tutti e tutte noi a fare in modo che la piaga della criminalità organizzata possa trovare nelle leggi dello Stato, ma anche e soprattutto nella testimonianza civile delle persone in prima linea, una soluzione, fornendo una via di salvezza salvezza al nostro Paese dal crimine organizzato, per la riaffermazione della legalità dello Stato e della piena costituzionalità della vita di tutti i nostri concittadini e concittadine, anche quelli che vivono nelle zone maggiormente colpite da questa piaga.

Avverto che la 5a Commissione ha espresso sul testo del disegno di legge proposto dalla Commissione giustizia un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1. Peraltro, come già rilevato dal senatore Tonini nel corso della seduta della 5a Commissione permanente del 13 dicembre scorso, l'emendamento del relatore 1.1, che incide proprio sul comma 2 dell'articolo 1, ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati sul quale la stessa Commissione bilancio aveva espresso un parere integralmente non ostativo.

Presidente, confermo quanto da lei detto: è evidente che il nostro parere contrario sul comma deve intendersi come un parere di nulla osta condizionato all'approvazione dell'emendamento. Ove approvato l'emendamento, ovviamente, le obiezioni cadrebbero. Alla luce di quanto illustrato dal senatore Tonini, l'approvazione dell'emendamento 1.1 è necessaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passiamo all'esame

Grazie Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame mira a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991. Il disegno di legge dà seguito alle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella sua relazione sul sistema di di protezione dei testimoni di giustizia, presentata nell'ottobre 2014. Va preliminarmente ricordato che la legge n. 45 del 2001, riformando appunto la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collaboratori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del testimone di giustizia, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai cosiddetti pentiti, normalmente estranea al circuito criminale. Prima del 2001, infatti, il trattamento del testimone, nella prassi, era indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta per quanto riguarda sia la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione, sia il trattamento. La disciplina sui testimoni è stata poi integrata per via regolamentare: soprattutto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 161 dell'aprile 2004, nonostante il carattere di normativa secondaria, ha svolto un fondamentale ruolo Grazie di natura premiale - in cambio di benefici di varia natura (penali, processuali, penitenziari ed economici), per sé e per i propri familiari - nonché di protezione fisica, per sé e per le proprie famiglie. I cosiddetti pentiti sottoscrivono un contratto con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono. I testimoni di giustizia, invece, sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con la criminalità e decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto reato, spesso rispondendo ad un dovere civico che nel nostro Paese sta sempre più venendo Godono per questo di una protezione da parte dello Stato che, come per i pentiti, spazia dalle misure di tutela fisica allargate ai familiari a quelle economiche e di reinserimento sociolavorativo. La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui identità sociale è più sfumata: imprenditori stanchi di pagare il pizzo, soggetti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere

un'insufficiente definizione dello *status* di testimone; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione, che comporta il suo sradicamento dal luogo di residenza; il il *deficit* informativo sui suoi diritti e i suoi doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento sociolavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalle mancanza di referenti certi; infine, la mancata previsione di un termine di durata delle misure. Le numerose problematiche applicative, come si legge anche nella relazione illustrativa della proposta di legge, hanno fatto ritenere che il decreto-legge n. 8 del 1991 non potesse più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che invece occorresse una specifica legge destinata a tale peculiare figura. Tra le novità previste da questa riforma, si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e la gradualità delle misure (e, in tale ambito, è data preferenza all'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato con programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito; di reddito; l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone. C'è poi l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità. Infine, è prevista l'introduzione di un termine di durata massima delle misure. Quella che ci preme segnalare in questa sede è una delle novità più significative introdotte con questa proposta di legge che, come ho detto prima e ripeto, Grazie di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali. 2. Il

tra questi e la Commissione centrale per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela. Mi avvio alle conclusioni, cari colleghi, per dire che il Gruppo Lega Nord e Autonomie condivide questa proposta di legge che vuole riconoscere il testimone di giustizia come il cittadino che adempie ad un dovere civico che garantisce e contribuisce con le proprie deposizioni all'individuazione di responsabilità nell'ambito della criminalità organizzata e non solo e che dunque, versando in una situazione di rischio e talvolta di elevato pericolo,

discusso in Aula e trovasse lo spazio per essere approvato prima della fine della legislatura, perché gli riconosciamo un'enorme, gigantesca importanza politica e sociale per combattere la criminalità organizzata. In effetti credo che l'opinione pubblica facesse fatica a capire la serie, magari anche eccessiva, di privilegi dati ai cosiddetti pentiti, ai collaboratori di giustizia, che non sempre hanno dimostrato di meritare il trattamento privilegiato che lo Stato ha rivolto loro: stiamo parlando anche di personaggi che hanno alle spalle decine e decine di omicidi,

che pesavano sul sentimento popolare di giustizia. I testimoni di giustizia sono tutt'altra cosa, siamo proprio sul versante opposto: parliamo di persone perbene, parliamo di persone perbene, incensurate e che mettono a rischio la loro vita, la loro incolumità, i loro beni e la pace sociale, anche della loro famiglia, perché hanno il coraggio di essere testimoni contro la criminalità organizzata.

agente di commercio, mentre si trovava a viaggiare lungo la statale Canicattì-Agrigento si trovò ad assistere all'omicidio del giudice Livatino (poi divenuto famoso come il giudice ragazzino) e non esitò, appena giunto a destinazione, a chiamare le forze dell'ordine e a dare un contributo fondamentale per l'identificazione e la condanna degli assassini. In più occasioni il signor Nava ha avuto poi modo di affermare di non essere un eroe e di non sentirsi tale. Eppure, il suo gesto ha determinato lo stravolgimento della sua vita. Da quel momento egli ha vissuto la sua vita nel contesto di un sistema di protezione che vedeva i suoi primi passi e che era stato, in realtà, pensato e strutturato per i cosiddetti collaboratori di giustizia. Sennonché, i collaboratori di giustizia, ai quali il legislatore ha riservato molta più attenzione, sono e devono essere, per poter fornire un contributo investigativo utile efferati criminali che, nella maggior parte dei casi, decidono di rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie al solo scopo di sfuggire alle severe pene che, di fatto, meriterebbero. Quindi, con soddisfazione, fermo restando il rammarico per il ritardo, licenziamo oggi il primo intervento normativo organico pensato espressamente per i testimoni di giustizia, che tenga conto della loro specificità e della necessità di evitare, anche a costo di un maggiore impegno economico e protettivo dello Stato, e salvo casi eccezionali, lo sradicamento dal territorio e l'interruzione delle attività professionali e imprenditoriali del testimone. Certo, vi è il rischio che taluno, per convenienza economica, mitomania o altro (lo dico con cognizione di causa, per essere un fatto del genere avvenuto proprio nella mia città di Torre del Greco), voglia o possa simulare di essere stato vittima di gravi reati o di avere assistito alla loro la legge oggi licenziamo ha disegnato una commissione centrale, composta da soggetti qualificati, cui vengono affidate le indagini, gli esami e la valutazione della veridicità dei fatti che denuncia il testimone, credo quindi che detto rischio

decorsi i termini della *vacatio legis*, diventare legge nel nostro Paese. Abbiamo dato un contributo in questa direzione e siamo orgogliosi di aver lavorato insieme a tutti i colleghi. Questo è oggi un successo di questo Senato, nel momento in cui il provvedimento passa all'unanimità, così come all'unanimità sono stati bocciati gli emendamenti. Anticipo il voto del mio Gruppo, favorevole a questo testo. Con soddisfazione, questo stralcio di fine legislatura veramente acquista un significato valido nell'interesse del nostro del nostro Paese e nella lotta alla criminalità organizzata. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Papa Francesco, quando ci ha ricevuti come Commissione antimafia all'udienza speciale, il 19 settembre, in Vaticano, disse: «Non si può dimenticare che la lotta alle mafie passa attraverso la tutela e la valorizzazione dei testimoni di giustizia, persone che si espongono a gravi rischi scegliendo di denunciare le violenze di cui sono state testimoni. Va trovata una via che permetta a una persona pulita di uscirne senza subire vendette e ritorsioni». Finalmente allora arriva nella nostra Aula la legge sulla protezione dei testimoni di giustizia. È ancora molta la confusione che fanno i cittadini fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. Come ha detto un testimone di giustizia, Rocco Mangiardi: «Ogni volta che qualcuno erroneamente o per incompetenza mi chiama collaboratore di giustizia, per chi come me non proviene da nessuna cosca mafiosa, bensì da una scelta di campo netta e precisa, è un vero pugno nello stomaco. Fosse per me, preferirei essere chiamato semplicemente per quello che in realtà mi sento da sempre di essere: cittadino responsabile». Uno degli obiettivi di questa legge è proprio deliberare uno statuto evitando di confondere le due figure sul piano giuridico, amministrativo e culturale. Il testimone di giustizia vive una condizione di grave pericolo, tanto che necessita di una protezione speciale rispetto alla protezione ordinaria. Nella gran parte dei casi il testimone, con il suo apporto, mette in crisi il modello mafioso e per questo corre gravi pericoli. Il testimone di giustizia deve avere, per essere tale, dei requisiti specifici: non deve avere benefici rispetto al reato che sta denunciando; non deve avere condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione a suo carico; la testimonianza deve essere attendibile e rilevante ai

Quel suicidio s'impose all'attenzione degli osservatori e del legislatore come già era successo per un'altra vicenda tipica degli ultimi venticinque anni, quella dell'ingegnere bergamasco che aveva assistito al barbaro assassinio di Rosario Livatino, e in seguito alla quale fu emanato il decreto-legge n. 8 del 1991. Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (convertito nella legge n. 82 del 1991) e dei sistemi di tutela ivi previsti, è poi venuta la tragica storia di Domenico Noviello, commerciante di Casal di Principe, ucciso ben sei anni dopo il termine del programma di protezione.

a causa dell'ingerimento di dieci bicchieri di acido muriatico. E poi ancora la terribile vicenda del costruttore Giuseppe Masciari, del commerciante Tiberio Bentivoglio di Reggio Calabria e di molti altri. Le storie dei testimoni in pericolo non sono *film* in prima visione, come quello con Harrison Ford, «Il testimone»; sono percorsi di rovina, di abbandono, di tradimento sottile e di burocratica solitudine. La proposta di legge della Camera n. 3500 costituisce sicuramente un passo in avanti, ma altri ne dovranno essere fatti. Il vero problema dei testimoni di giustizia è la pubblicità della loro identità. Questa pubblicità sembrerebbe necessitata dalla regola processuale della formazione della prova in contradditorio. In realtà non è così. L'articolo 111, quinto comma, della Costituzione prevede che a questa regola si possa derogare per motivi di provata condotta illecita. Sicché Sicché nella proposta che oggi convintamente ci accingiamo ad approvare si poteva fare una scelta più coraggiosa, cioè stabilire che il caso dei testimoni di mafia è sicuramente di comprovata condotta illecita e quindi escludere la deposizione a processo dei testimoni di giustizia,

Grazie

un complesso e lungo lavoro della Commissione antimafia tutta (desidero sottolineare questo), coadiuvata dal quinto comitato coordinato dall'onorevole Mattiello. Sono stati auditi molti testimoni di giustizia, sono state raccolte le loro storie: come vivono la loro condizione, come sono stati aiutati dallo Stato. Naturalmente sono state audite anche le istituzioni, dalla magistratura alla Commissione centrale, ai vari attori del sistema che sovrintendono ai loro bisogni. Dall'analisi delle situazioni riscontrate sono emerse numerose criticità, espresse nella relazione votata all'unanimità il 21 Tenendo conto delle considerazioni riportate dalla relazione, la Commissione antimafia ha predisposto un disegno di legge che è stato presentato alla Camera a prima firma dell'onorevole Bindi ed al Senato a mia prima firma (l'Atto Senato 2176). Credo che oggi segniamo un punto molto importante nella civiltà giuridica del nostro Paese. Non era possibile continuare a disciplinare con la stessa legge, ispirandoci tutto sommato agli stessi principi e alle stesse modalità, persone che, per quanto siano entrambe preziose per la lotta alla criminalità organizzata, sono profondamente diverse. I collaboratori di giustizia sono persone che si sono macchiate anche di delitti efferati e hanno fatto parte integrante delle organizzazioni mafiose; i testimoni di giustizia sono cittadini normali, che hanno subito la violenza delle mafie o che hanno assistito alle estorsioni, ai ricatti, ai patti corruttivi delle mafie, li hanno denunciati e si sono recati nelle aule giudiziarie ad indicare i colpevoli di quei reati. Penso che anche solo i numeri siano indicativi: non era possibile che nella stessa legge e con gli stessi sistemi di protezione noi garantissimo i collaboratori di giustizia, che sono 1.277 con 4.915 familiari, e i testimoni, che sono 78, e i 255 loro familiari. Questa legge dà loro uno statuto autonomo e una dignità nel nostro sistema che essi meritavano, che meritano, e che attendono da troppo tempo. Credo che dobbiamo sottolineare questo aspetto con molta forza. Il secondo aspetto del disegno di legge in discussione è il principio della personalizzazione: ciascun testimone di giustizia e la sua famiglia sono persone con la loro peculiarità, la loro originalità, la loro storia; non si poteva pretendere che per ciascuno di loro venissero applicate misure standardizzate. Il testimone di giustizia non può subire e continuare a subire quello che ha subito in questi anni, come lo sradicamento dal proprio territorio, il cambiamento del nome per sé e per la propria famiglia, l'abbandono del proprio lavoro, del proprio territorio, della propria impresa. Non sono loro che devono abbandonare i loro territori, ma sono le mafie che, dalla loro testimonianza nel loro territorio, devono essere cacciate, laddove hanno fatto da padroni, hanno ucciso, hanno corrotto, hanno ricattato. La normalità d'ora in poi sarà questa: un testimone di giustizia dovrà essere assicurato (lui e la sua famiglia) da un sistema di sicurezze a casa propria, dove potrà continuare il proprio lavoro e, se è un imprenditore, la propria impresa. Ritengo che abbiamo fatto bene anche a considerare residuale l'assunzione nella pubblica amministrazione, per ciascun testimone di giustizia o referente che lo accompagna, anche nell'autorizzazione delle risorse, che non sono state poche in questi anni, ma che spesso non hanno fruttato, proprio proprio perché lo stesso testimone di giustizia ha dovuto fare i conti con turbamenti profondi della sua vita, del suo equilibrio e della sua famiglia. Altro punto qualificante è l'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione ed anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale. Concludo signora Presidente, con le stesse parole pronunciate dalla presidente Bindi alla Camera, come segno di continuità della Commissione antimafia di Camera-Senato: «Dedichiamo questa legge a ciascun testimone di giustizia, speriamo che sia un po' riparatrice di tutte le sofferenze di questi anni, per ciascuno di loro e per le proprie famiglie. Ma non sentiamoci sollevati nella nostra coscienza di cittadini, perché di testimoni di giustizia potremo fare a meno il giorno nel quale ciascuno di noi sarà un testimone di giustizia e ciascuno di noi si sentirà un presidio di legalità e di cittadinanza contro ogni forma di criminalità.». *(Applausi

È con grande soddisfazione che arriviamo oggi all'approvazione finale di questo importantissimo provvedimento. Per molti anni, signora Presidente, colleghi, il coraggio e il senso civico di tanti uomini e donne di questo Paese non sono stati ripagati, come sarebbe stato giusto fare. Non sono stati protetti, come sarebbe stato giusto fare. Imprenditori che hanno denunciato e semplici cittadini che hanno assistito a un reato sono spesso rimasti soli e a volte trattati, dal senso comune, come pentiti, proprio perché la legge regolamentava la loro collaborazione allo stesso modo. Hanno vissuto con pochi euro al mese. Alcuni con pacchi alimentari della Caritas, altri hanno dovuto affrontare processi senza le adeguate misure di sicurezza. Hanno vissuto e vivono nella paura per sé e per i propri familiari. Tutte le audizioni e il lavoro svolto in Commissione antimafia, che ha consentito di approvare, nell'ottobre del 2014, una relazione sulla revisione del sistema di protezione per i testimoni di giustizia, ha reso un quadro chiaro che ci ha dato - credo - gli elementi per arrivare a una profonda revisione del sistema e a questo disegno di legge. Il decreto-legge n. 8 del 1991, con cui, a partire dal 2001, oltre ai collaboratori veniva normato il trattamento dei testimoni, come si è visto da questa relazione e da tutto quello che è accaduto nel quadro che ci è stato dato degli ultimi anni, si è dimostrato assolutamente insufficiente, se non addirittura ingiusto. I testimoni hanno pagato spesso con l'isolamento geografico e sociale, perdendo il proprio lavoro e a volte le proprie case. Hanno assistito a disparità di trattamento economico tra loro, a una burocrazia farraginosa e dannosa, che spesso (basti guardare a molte testimonianze) li ha fatti pentire addirittura di aver denunciato. Eppure le loro testimonianze sono state fondamentali per la giustizia italiana. Sono state fondamentali per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Grazie a loro negli ultimi anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata e alla criminalità in generale. Hanno fatto del senso della giustizia una loro ragione di vita e non sono stati, appunto, adeguatamente protetti. Il loro aiuto è stato fondamentale e, oltre a ringraziarli per questo, possiamo finalmente, con questa proposta di legge che modifica il decreto-legge del 1991 e alcune parti del codice penale, definire finalmente una disciplina organica specifica. Per questo motivo, come senatori di Sinistra Italiana-Libertà e Uguaglianza, voteremo a favore di questo provvedimento, come abbiamo votato a favore di tutti i provvedimenti che sono stati messi a disposizione del contrasto del fenomeno mafioso. Certamente eravamo in forte ritardo, ma finalmente, anche nelle ultime ore di questa legislatura, riusciamo a colmare questo vuoto che ci portavamo avanti da molti anni. Certo non è un provvedimento perfetto, lo sappiamo bene, anche perché ancora una volta le risorse finanziarie non sono moltissime. Quindi, da questo punto di vista, bisogna riconoscere

sia nell'individuazione della definizione del testimone di giustizia, sia, essenzialmente, nel procedimento per applicare le misure di tutela. misure di tutela. Tali misure sono state individuate correttamente, anche tenendo conto della necessità di garantire il reinserimento sociale del testimone di giustizia, non solo con un contributo economico, ma anche con un aiuto all'attività lavorativa. La valutazione complessiva è certamente positiva, da un lato per il contributo che i testimoni di giustizia danno all'amministrazione della giustizia e all'accertamento delle responsabilità di coloro che si macchiano di delitti gravi e, dall'altro, perché abbiamo la necessità di garantire

esame sia un provvedimento complessivamente positivo, che si aspettava da anni, e che quindi voteremo con soddisfazione.

un impegno riconoscente verso chi mette a repentaglio la propria sicurezza per combattere il crimine e favorire la legalità. La sicurezza dei

scegliere di fare il testimone di giustizia non voglia dire una penalizzazione eccessiva, non voglia dire essere sradicato del proprio comune, dalla propria vita, dal proprio ambiente. Garantiamo reddito, casa e lavoro e, soprattutto, mettiamo in campo procedure chiare, trasparenti, efficaci ed efficienti per dare garanzie a chi decide di testimoniare. Diamo certezza dei tempi. La legge dà strumenti per percorsi personalizzati, che tengano conto dei rischi che corre il testimone e tiene conto del contesto familiare. [**Presidenza del presidente perché troppe persone, in questi anni, troppi testimoni di giustizia hanno subìto troppi disagi per aver scelto di stare della parte dello Stato. Non deve più succedere e questo provvedimento va in questa direzione, nella direzione giusta: sostenere i testimoni, stabilire non solo il principio ma soprattutto prevedere misure concrete. A chi testimonia va riconosciuto il A chi testimonia va riconosciuto il ruolo che ha svolto per sconfiggere le organizzazioni criminali. Questo è il senso di questa legge. Fatemi dire che è l'ennesima legge costruita in un dialogo tra Parlamento, Commissione antimafia, associazioni e Governo. Con questo disegno di legge - e ci tenevamo a terminarne l'*iter* prima della fine della legislatura - concludiamo un percorso che ha prodotto, in questa legislatura, uno straordinario numero di norme che hanno migliorato la legislazione antimafia, dato più forza allo Stato contro le cosche, dato più strumenti alle Forze dell'ordine e alla magistratura per combattere le mafie. Fatemi elencare alcuni dei provvedimenti. Sono 24 i provvedimenti importanti (come attestano Avviso Pubblico e Libera) che ha fatto questo Parlamento: sull'autoriciclaggio, a quelle sugli ecoreati, alla legge sul caporalato, alla legge anticorruzione, alla riforma del codice antimafia e dei beni confiscati. Oggi votiamo un provvedimento importante e credo sia un bel messaggio, ancora più forte se tutto il Parlamento, come mi pare sarà, oggi lo voterà Daremo un ulteriore segnale, tutti insieme, di un impegno comune di tutte le istituzioni di questo Paese contro le mafie. Questo è un messaggio che ha attraversato tutta la legislatura.

Signor Presidente, colleghi, illustro l'Atto Senato 2719 già approvato alla Camera all'unanimità. Questo testo si rende necessario per garantire ulteriori tutele agli orfani di femminicidio o comunque a tutti gli orfani di crimini domestici. Nel corso dei lavori di Commissione è stato rilevato come questi minori orfani normalmente, purtroppo, di uxoricidio siano di fatto bambini che subiscono un doppio trauma e nell'istante maledetto nel quale, nella maggioranza dei casi, la loro madre viene uccisa dall'uomo che questa donna amava, spesso dal padre dei bambini o comunque dall'uomo con cui questa donna conviveva, dall'altro *partner* della coppia dell'unione civile, dal convivente, questi bambini perdono di fatto entrambe le figure genitoriali di riferimento. In quel maledetto istante, questi bambini si trovano immediatamente soli, perdendo le due figure genitoriali con le quali erano cresciuti fino a quel momento. Di fatto, questi minori non sono equiparabili agli orfani di altri omicidi volontari, agli orfani di incidenti sul lavoro, agli orfani di crimini violenti

se ne ritrovano comunque vivo, accudente ed accogliente un altro, mentre l'orfano di crimini domestici, nel perdere la madre, automaticamente perde il padre che viene condannato all'ergastolo e comunque viene allontanato dalla vita famigliare. Molto spesso questi bambini - ed è su questo che lavora molto bene questo testo - si sono trovati già a vivere in una condizione di violenza assistita, a coesistere con questa abnorme violenza domestica e ineluttabilmente hanno ritenuto che quella fosse la loro normalità. Questi piccoli crescono in condizioni di fortissimo disagio psicologico, in una condizione nella quale ritengono che la violenza sia normale, abituale, e quindi è necessario, con questo provvedimento,

l'articolo 3, molto, importante sul sequestro conservativo dei beni dell'uxoricida, a garanzia del risarcimento dei danni civili che saranno poi liquidati nel corso del procedimento a vantaggio dei minori; l'articolo 4, che prevede una provvisionale, quindi una somma di denaro che viene

che prevede l'indegnità a succedere, con la finalità di rendere automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio: ci troviamo spesso nel caso abnorme in l'uxoricida non solo è erede legittimo in quanto legittimato in primo grado sui beni della donna che ha ucciso, ma addirittura può fruire della pensione di reversibilità . Ebbene su questo si interviene con una sospensione della fin dal momento dell'indagine. Questa disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, perché

orfani per vittime di incidenti sul lavoro. L'articolo 7 esclude dal diritto alla pensione di reversibilità, quindi è direttamente collegato a quanto abbiamo detto in precedenza. L'articolo 8 si riferisce a tutto quel lavoro sociale inclusivo e protettivo che bisogna costruire intorno agli orfani di crimini domestici. Si tratta di assistenza, consulenza, sostegno,

li ritiene soggetti che vanno gradualmente verso una vittimizzazione secondaria. Frenare e diminuire il livello di vittimizzazione secondaria è lo scopo dell'articolo 8, con cui si costruisce una rete sociale intorno a questi bambini.

l'articolo più importante resta il 10, in tema di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. Si rivolge un'attenzione fortissima alla continuità degli affetti e si snelliscono tutte quelle norme su affido e adozione che rendono questi istituti

a fine legislatura sentiamo tutti la necessità di approvare in via definitiva quei provvedimenti per cui non esiste più la possibilità di un ulteriore passaggio parlamentare. La Camera ha deciso di indicare, come beneficiari delle nuove misure, quei figli minori o maggiorenni non autosufficienti

usiamo un termine neutro, ma sappiamo che, nella grandissima parte dei casi, stiamo parlando della genitrice, della madre - nel caso in cui la madre o, in casi più limitati, il padre vengano uccisi per mano del proprio marito o, eventualmente, della propria *partner* in unione civile o di persona che abbia intessuto con il genitore una relazione affettiva e una stabile

Ma non dobbiamo dimenticare che, quando parliamo di femminicidio, in tanti casi parliamo dell'uccisione di donne da parte di persone che non sono il marito, il *partner* stabile o un *ex* convivente ma, magari, persone che hanno avuto un rapporto semplicemente hanno avuto un rapporto solo nella loro fantasia malata, unidirezionale, non fondato su una vera comunione o addirittura su una convivenza. Sarebbe stata molto importante una modifica di questo genere nel testo e sarà molto importante che, nell'interpretazione di questa legge, e poi - chissà -

casi, che poi sono fatti di cronaca conosciuti e *-* ahimè - tristementefortemente ripetuti in questo Paese. Nei mesi scorsi, grazie anche all'iniziativa

che non bastano l'azione penale e i risarcimenti. Occorre, per combattere questa piaga, un intervento forte e importante sul tema della relazione tra i generi. Esiste una questione maschile nel nostro Paese che non viene adeguatamente affrontata; esiste il tema di un rapporto tra uomini e donne che troppo spesso produce relazioni malate. Credo che sia molto importante che, a partire dall'azione culturale, dalle scuole, dall'educazione, riusciamo a intervenire su questo tema, facendo in modo che il rapporto tra le persone e, in particolare, il rapporto tra i generi riacquisti una dimensione fondata sul rispetto reciproco e mai sul senso di possesso o addirittura sull'atteggiamento violento. *(Applausi

Dal 2000 a oggi 1.628 sono gli orfani di madre uccisa nelle liti domestiche, in famiglia. Nel 2015 ci sono stati 118 orfani in più rispetto al 2014. Dispiace che il ritardo, spesso invocato da alcune parti politiche e imputato al mio Gruppo, sia stato strumentalizzato, su un argomento come questo, per attacchi vergognosi. Infatti, nel testo che ci è giunto dalla Camera si sono manifestati problemi legislativi che richiedevano un approfondimento. Purtroppo però, in questi anni, troppo spesso abbiamo assistito a leggi licenziate in modo frettoloso, che daranno luogo a contenziosi. Basti considerare l'ultima, sulle disposizioni anticipate di trattamento:

saranno modifiche e che si aprirà all'obiezione di coscienza». Ora, sempre per motivi elettorali, probabilmente, si è attaccata alla posizione di Forza Italia. Vorrei ricordare che

nel 2017, con la riforma del codice penale, addirittura era stata introdotta la possibilità di estinguere il reato pagando. Il tribunale di Torino aveva dato un indennizzo Finalmente, da poco, ma con molto ritardo, il Ministro delle pari opportunità, dopo molte promesse, ha fatto sì che questa possibilità potesse essere cancellata.

credo che il fatto di dire che ci sono pochi soldi non sia una giustificazione per distinguere tra orfani di serie A e di serie B. La nostra volontà di arrivare a una legge condivisa si è dimostrata fin da quando nella discussione alla Camera dei deputati

Questi bambini rivivono certamente ogni istante un fatto che però si vuole quasi far loro dimenticare. Della lettura di un libro che mi ha colpita moltissimo, «Orfani speciali», ricordo in particolare

viene completamente cancellata, modificata, esattamente come si è detto poco fa per i testimoni di i testimoni di giustizia che, nell'arco di poche ore, vengono strappati a tutto il loro ambiente e l'ambiente è fatto di molte cose (di casa, di cose, di amici, di persone, di abitudini e di tranquillità). Questi bambini

di psicoterapia, tra famiglia affidataria e scuola. La stessa famiglia affidataria vive certamente una rivoluzione nella propria casa,

e questi bambini hanno bisogno di rete, di competenze psicologiche, sociali, giuridiche, politiche e di servizi sul territorio e, a questo proposito, gli articoli 8 e 9 specificano le tutele che si vogliono dare. Mi auguro davvero che, al di là delle speculazioni politiche, che vengono sfruttate forse per altri fini e non per la tragedia di cui si sta parlando, si possa arrivare a una serena discussione e approvazione dei nostri emendamenti per poter concordare un testo veramente utile, che sia qualcosa di importante per far sentire a quei bambini che lo Stato esiste. *(Applausi

l'assassino deve essere una persona sposata, anche se legalmente separata o divorziata; deve essere una parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o una persona che è

L'assassino non faceva parte di una unione civile. L'assassino non ha mai avuto una stabile convivenza affettiva. Anzi, era un molestatore che voleva avere la donna e, essendo stato rifiutato, l'ha ammazzata. Vogliamo fare un altro esempio? una persona che è stata sposata, poi si è separata e da vent'anni si è fatta un'altra famiglia e vive con un'altra donna. Mettiamo che vent'anni dopo, per una serie di questioni, magari di interesse, uccida o il padre o la madre dei bambini.

perché chi ha causato l'omicidio stradale non è sposato, né è parte di unione civile, né ha avuto in passato una relazione stabile con una delle due persone facenti parte

compiuto da un molestatore o da qualcuno che faceva parte della famiglia o a causa di un omicidio stradale o compiuto da un rapinatore rimane orfano, gli viene garantita l'assistenza legale perché è rimasto traumaticamente privato del padre e della madre. non è così, perché qui il soggetto della legge non è l'orfano: il soggetto della legge sono le persone sposate o separate sono quelle in unioni civili, anche se cessate; sono quelle che hanno avuto una relazione stabile. Quindi, noi andiamo ad assistere bambini che, pur nella tragedia che hanno vissuto, hanno ancora uno dei genitori in vita, che li può assistere, e non andiamo ad assistere, invece, bambini che rimangono orfani di padre e di madre essendo stati sì uccisi,

una volta che gli viene tolta la casa e gli viene confiscato tutto, i bambini minori di costui che tipo di tutela hanno? Colleghi, se parliamo di omicidio domestico perché si tratta di persone conviventi,

anche ai bambini che rimangono orfani, vittime di omicidi - sto parlando di quelli che tecnicamente il codice definisce omicidi - diamo loro lo stesso trattamento che diamo agli altri bambini.

reca «disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici». Il crimine molte volte non è domestico e non c'entra affatto con la convivenza di uomini e donne della loro famiglia: non è un crimine familiare nell'ambito della famiglia; della famiglia; gli orfani, in qualche caso sono orfani, in qualche altro caso non sono affatto orfani, perché rimane loro un genitore per assisterli (magari, nell'unione civile, è il genitore biologico, cioè il vero padre, perché la madre è da un'altra parte con chi non c'entra niente, quindi gli rimane un genitore),

quelli sposati, quelli delle unioni civili, quelli che hanno avuto una relazione sentimentale stabile in passato. Ma non si parte dal punto di vista dei bambini: i bambini che sono rimasti orfani a seguito di omicidio hanno diritto a una tutela legale, perché hanno lo stesso trauma e gli stessi problemi, le stesse tragedie psicologiche, vivono lo stesso dramma. Perché non devono essere trattati tutti allo stesso modo? Non c'è l'articolo 3 della Costituzione? Non c'è un sentimento popolare che si indigna pensando che un bambino non abbia il supporto delle istituzioni nel momento in cui traumaticamente si vede eliminare i genitori, e il contesto familiare in cui vive e da cui viene allontanato?

Viceversa, se ammazzano sia il padre che la madre ma l'assassino non ha avuto una relazione stabile con uno dei due, il bambino rimane totalmente da solo, senza nessuna tutela. Capisco che la casistica va messa in fila, ma quando vedremo gli emendamenti vi accorgerete che le cose sono esattamente così. Capisco che ci sono le questioni di bilancio. Si dice che dobbiamo dare un segnale.

E daremmo assistenza legale a tutti quelli che voi dite devono avere assistenza legale, perché non ho nulla da obiettare a quanto la relatrice ha esposto. Mi sta benissimo, basta scriverlo,

dovrebbe essere fissato il sacrosanto diritto per tutti bambini che a causa di un omicidio perdono i genitori. La collega ha parlato anche dei poliziotti e dei carabinieri: certo, quando un poliziotto o un carabiniere viene ucciso in servizio

calpestando i diritti dei bambini e l'articolo 3 della Costituzione, nonché creando una situazione insostenibile. Se volessi fare polemica, chiederei

ad avere assistenza, soltanto perché il molestatore non è mai stato sposato o non è mai riuscito ad avere una relazione stabile con quella donna (anzi la molestava perché la voleva e lei lo rifiutava). In quei casi i bambini hanno assistenza? No, mancano i presupposti: i genitori non erano sposati,

orfani, in qualsiasi situazione ciò accada, a causa di un omicidio, in maniera traumatica, e non sia invece l'ennesimo manifesto ideologico da sbandierare in giro per il Paese

oltre a gettare nello sgomento la famiglia e gli amici, ha fatto venir meno un'importante figura di riferimento per il mondo politico e istituzionale. I fiori sul posto da lui occupato dimostrano che lui è e rimarrà ancora con noi. Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare e istituzionale, Altero Matteoli ha ricoperto tante cariche che saranno certamente illustrate, ma a me premeva ricordare che è stato un uomo profondamente legato ai valori dell'istituzione parlamentare. Indiscutibile la sua abilità nel perseguire soluzioni di mediazione politica, sostenuta da una profonda capacità di ascolto e del rispetto delle posizioni altrui. Con lui perdiamo, come unanimemente riconosciuto dagli amici ma anche dagli avversari, non solo un uomo politico di alto spessore ma anche un parlamentare leale, dal tratto affabile e cortese, che abbiamo avuto il privilegio di notare - almeno io personalmente, essendo questa la mia unica esperienza parlamentare - anche in questa legislatura. Tutte doti che gli hanno permesso, peraltro, di condurre in questi anni, con grande equilibrio ed autorevolezza, le sedute della Commissione lavori pubblici. Desidero pertanto esprimere il commosso cordoglio del Senato della Repubblica alla famiglia di Altero Matteoli, nonché agli amici alla comunità politica, colpita dalla scomparsa di un uomo delle istituzioni e di un importante esponente della destra italiana. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto alla famiglia di Altero, la famiglia del presidente Matteoli. Sono seduti nelle tribune la moglie Ginevra e i figli Federico e Federica. *(Generali

un saluto a nome di tutti i senatori di Forza Italia e ringrazio anche gli altri Gruppi. Vorrei spendere alcune parole più per l'amico Altero che per il politico, per l'uomo delle istituzioni che tutti, in quest'Aula ma anche fuori, hanno avuto modo di conoscere, di apprezzare e stimare. Gli attestati di stima e di affetto di questi giorni sono stati veramente tanti, a partire dai tanti colleghi senatori di tutti gli schieramenti, di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in quest'Aula. Lascerò poi la parola al vice presidente Gasparri che ha condiviso con Altero tanti anni di battaglie politiche, di militanza di partito, di amicizia e di vita, ma se il legame che ho avuto modo di stringere con Altero è stato sicuramente più recente di quello che lo ha legato al presidente Gasparri non è stato però meno intenso. I nostri percorsi politici ci hanno consentito di incontrarci tantissime volte nel corso degli ultimi vent'anni. Siamo stati anche al Governo insieme, ma è stata soprattutto la condivisione di questi banchi al Senato che ci ha consentito di stringere ancora di più un rapporto di amicizia straordinario. Un rapporto che è andato oltre all'appartenenza allo stesso partito politico e allo stesso Gruppo parlamentare. Io, colleghi, quel 18 dicembre ho perso un amico, un caro amico, un uomo che stimavo, cui ho voluto molto bene. Un uomo di cui ascoltavo i consigli, con cui ho condiviso opinioni, riflessioni, con il quale mi sono sempre consultato prima di assumere decisioni politiche e con il quale ho amato fare politica, perché la passione politica per Altero era indiscutibile ed era capace di trasmetterla anche nei momenti in cui noi perdevamo l'entusiasmo, la sentivamo o la vedevamo svilita. Di Altero ho apprezzato sempre la forza, la determinazione, ma anche e soprattutto - lo hanno detto in tanti - la straordinaria capacità di mediazione. Avrei voluto soffermarmi solo sulle qualità umane di Altero, ma non posso non rilevare, al fondo di questo mio breve intervento, che la politica italiana ha perso in lui un uomo di grande, straordinaria esperienza, di grande e straordinario valore, di grande e straordinaria qualità. La perdita di Altero, del presidente Matteoli, lascia in tutti noi e in me un vuoto veramente incolmabile.

in maniera improvvisa e dolorosa, non solo chi come me ed altri ha condiviso con Altero decenni - perché di questo si tratta - di vita comune, ma direi più vastamente la comunità politica, il mondo delle istituzioni, come l'abbiamo visto anche in queste ore, salutando con affetto i familiari, i figli e Ginevra (che Altero ha conosciuto in Parlamento, perché Ginevra era una giornalista parlamentare, quindi anche questo legame è nato nella pratica e nella frequentazione dei luoghi della democrazia

sono dei professionisti della politica quelli che ad un certo punto della vita lasciano un'altra attività e vanno a fare il candidato momentaneo. Altero Matteoli è stato un militante politico, come tanti altri di noi lo sono in quest'Aula e rivendicano con orgoglio questa definizione della militanza, dell'appartenenza ad uno schieramento, della testimonianza delle idee: oggi non so se sia intesa come lo era un tempo. Altero non amava la retorica; lo avete conosciuto, la sua sobrietà e la sua concretezza ci impongono di evitare discorsi di maniera, ma cerco invece di dare spazio a poche considerazioni sentite. Altero è stato un uomo d'azione, nei nostri partiti, nella realtà del centrodestra, si è sempre occupato di organizzazione, di trovare intese, di preparare elezioni; delle cose concrete della politica, perché poi tutti parlano ma ci vuole qualcuno che organizzi gli strumenti per rappresentare le idee. Tuttavia,

di pensiero, quindi un po' pensiero e un po' azione, una dicotomia che ci porta al Risorgimento, cui anche tanti segni di quest'Aula ci richiamano. Riviste, fondazione, convegni, dibattiti: Altero non è stato solo un infaticabile organizzatore, ma anche un promotore di pensiero capace di ascolto e di affermazioni, e anche nelle ultime settimane con la sua fondazione, oltre con l'azione politica in Forza Italia, ha promosso incontri e convegni per tenere unite le fila di una coalizione (e tutti sappiamo, nei rispettivi ambiti, quanto sia difficile e quanto sia faticoso). Altero ha anche tenuto una linea coerente. A me è capitato di condividere questo percorso. Siamo venuti da una destra politica di cui siamo orgogliosi, quella del Movimento Sociale Italiano, della svolta di Fiuggi, di Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà (un grande schieramento, che poi si è frantumato), e oggi siamo in Forza Italia e con Berlusconi per ripercorrere un tentativo di unità del centrodestra. Quindi, c'è un filo in questo percorso, per creare un'Italia in cui dei grandi schieramenti - oggi, tutti con le loro fatiche - si possano democraticamente confrontare e contendersi pacificamente il governo del Paese. Anche in questi giorni, Altero ha testimoniato questa scelta. è stato l'unico Ministro in tutti i Governi guidati da Silvio Berlusconi (quello del 1994 e gli altri) e non perché scalpitasse dietro delle poltrone, ma perché la sua affidabilità e solidità

contano più della foga "rottamatrice": rottamiamo, sfasciamo, ricambiamo. Per carità, il ricambio fa parte della vita e della politica, ma l'esperienza e la saggezza, in epoche di frammentazione, sono risorse fondamentali, che Altero ha regalato a tutti noi. noi. A volte, una sentenza e una decisione ingiusta contano meno della reputazione che ha accompagnato Altero fino all'ultimo momento. Non voglio cedere alla commozione, ma ringrazio tutti coloro che gli stanno

La tragica e improvvisa scomparsa del senatore Altero Matteoli ha suscitato costernazione in tutto il mondo politico, ben oltre i confini del suo schieramento, a testimonianza di una personalità che ha saputo distinguersi per coerenza, passione e dedizione alle istituzioni. Ho detto oggi al figlio che deve essere orgoglioso dell'eredità di suo padre, perché ha sempre dimostrato, nella relazione con il Governo, una grande dedizione e un grande senso istituzionale.

a successo diverse riforme insieme. A dimostrazione di un senso istituzionale elevatissimo, non ha mai chiesto, per poter far procedere i provvedimenti, alcuna alcuna azione da parte del Governo, alcuno scambio politico: ha sempre chiesto e ottenuto di discutere nel merito delle questioni. Questo credo sia un esempio di grande lealtà, verso i bisogni dei cittadini, prima di tutto, perché noi facciamo le leggi per i cittadini. È entrato in Parlamento, alla Camera dei deputati, nel 1983, nelle fila del Movimento Sociale Italiano. Era un uomo di destra, quindi lontanissimo dalle mie idee; un uomo che era orgoglioso di saper prendere parte, ma posso dire che sapeva prendere parte senza essere di parte, senza essere sordo alle ragioni degli avversari. È questo un elemento di grande qualità, una testimonianza e un'eredità che credo dobbiamo raccogliere e conservare gelosamente in questa fase di transizione della Repubblica. Ha avuto al suo attivo un'intensa attività ministeriale: è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro dell'ambiente e di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nel Ministero che ho ora l'onore di presiedere ha avuto anche un ruolo importantissimo per la definizione del collegamento dell'Alta velocità Torino-Lione; in momenti molto difficili, ha siglato l'intesa con gli enti locali; ha saputo, in quegli anni, dare vita a un piano casa importante e rilevante per il Paese. L'attenzione agli enti locali si è rivelata anche quando ha deciso di accettare l'incarico a sindaco di Orbetello, tra il 2006 e il 2011, a dimostrazione di uno sguardo "strabico", che credo sia un'altra eredità importante che dovremmo tenere presente: lo "sguardo strabico" di chi sa guardare all'interesse nazionale, all'interesse del Paese, senza dimenticare il suo radicamento nella comunità locale, senza dimenticare l'intelligenza e la vicinanza alle comunità locali. Con Altero Matteoli viene a mancare una personalità politica che, in particolare nella stagione che si è aperta ormai più di vent'anni fa, ha contribuito con determinazione e - credo - scrupolo, al tentativo di modernizzare il nostro Paese e il nostro sistema, perché senza mai tradirne la natura parlamentare si indirizzasse verso una più matura capacità di governo e una più matura capacità decisionale. Rinnovo ai suoi familiari e a tutti noi, che gli abbiamo voluto bene, il sincero cordoglio e l'impegno a conservare vivo il ricordo della sua azione.

questa mattina abbiamo reso omaggio ad Altero Matteoli alla camera ardente qui in Senato e abbiamo salutato con commozione i suoi familiari, ai quali rinnovo il saluto, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico. Ora lo onoriamo qui in Aula. Io, se di lui dovessi dire una sola parola, direi che era un uomo e, se potessi aggiungere un solo aggettivo, direi che era un uomo serio. Con Altero Matteoli per tanti anni ci siamo osservati da lontano, dalle due sponde del Senato, lui dal centrodestra dell'emiciclo e io dal centrosinistra. Ma in Parlamento succede anche questo, che ci si osserva a distanza e, da lontano, ci si riconosce. Così è successo tra Altero Matteoli e me e credo di poter dire che, nonostante le distanze, ci conoscessimo bene e ci stimassimo vicendevolmente. Dicendo che era un uomo serio intendo dire non solo che ha diretto con molta serietà

È successo, lo ricordava prima il presidente Gasparri, quando Alleanza Nazionale, di cui era uno dei massimi dirigenti, si è fusa con Forza Italia nel Popolo della Libertà; è successo quando il Popolo della Libertà, per via della scissione, è tornato ad essere Forza Italia ed è successo ancora negli ultimi mesi, quando l'intero centrodestra è stato attraversato da un dibattito, in parte pre-elettorale, ma in parte consistente e anche di riorganizzazione politica. In tutte queste fasi, Altero Matteoli è rimasto se stesso. Anche se stare dall'altra parte dell'emiciclo, da dove lo seguivo, può spesso segnare una forte lontananza, ne ho sempre colto e rispettato la coerenza e l'equilibrio. Aveva un tratto tranquillo, qualche volta burbero e a volte quasi sereno. L'ho visto accendersi in Aula o nelle conversazioni che spesso facciamo durante i lavori solo quando il dibattito diventava politico: la sua natura prendeva allora il sopravvento, quasi non volesse lasciare dubbi sul suo essere schierato con la sua parte da cui stava. L'ho visto tornare sereno il 2 aprile 2015, quando ha preso la parola in Aula, non per difendersi dalle accuse sulla vicenda veneziana del MOSE, ma per chiedere che il Senato lo lasciasse giudicare dalla magistratura,

Dichiarava la sua innocenza e voleva che venisse dichiarata da una sentenza dei giudici, senza aggirare la giustizia, di cui pure denunciava gli errori, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Quel 2 aprile ho ascoltato con attenzione Altero Matteoli e ne ho ammirato la dignità, la compostezza e anche il decoro istituzionale. In un tempo in cui è frequente la tentazione di sfuggire il giudizio penale, Altero Matteoli, a testa alta e con voce ferma, quel giudizio lo chiedeva e quasi lo esigeva. Ripensando a quella mattina e alla sua richiesta di essere giudicato dalla magistratura come un comune cittadino, mi pento - e lo debbo dire oggi di non aver applaudito e di non averlo fatto solo per ragioni di schieramento, lui di destra e io di sinistra. Non l'ho fatto allora, ma lo faccio simbolicamente oggi, applaudendolo e salutandolo con tanta considerazione e rispetto, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico e mio personale.

per porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del senatore Altero Matteoli, Presidente della Commissione 8ª, lavori pubblici e comunicazioni, per quest'improvvisa e tragica perdita. Notoriamente, le rispettive posizioni politiche ci hanno visto su fronti contrapposti, ma vi è l'aspetto umano che va sempre rispettato. Possiamo senz'altro testimoniare che, in qualità di Presidente della Commissione, ha sempre onorato il suo ruolo istituzionale, con imparzialità verso tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione. Ciò ha sempre permesso di lavorare in modo organizzato e proficuo, seppur nella radicale differenza di opinioni sulle varie questioni sollevate nel corso della legislatura. A nome di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle, rinnovo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia.

a Presidente della 8a Commissione, dove vengo designato come Vice Presidente di opposizione. È evidente, quindi, il confronto nel merito dei principali provvedimenti, che è stato sempre netto e schietto. Ma è proprio questo il punto, che senza alcuna retorica definisco straordinario: l'assoluto rispetto istituzionale delle prerogative e responsabilità che derivano dalla carica svolta e l'esercizio libero delle idee e delle proposte che si ritengono di sostenere ed affermare. Questo si è visto attraverso la qualità e quantità del lavoro svolto dalla 8a Commissione, spesso unitario e schietto, autonomo nel rapporto con il Governo. È stato un determinato sostenitore della realizzazione, da circa venti anni, dell'autostrada tirrenica; io sono stato, e resto, fieramente contrario a questo progetto, ma una cosa la voglio assolutamente dire: non ha mai esercitato in maniera impropria il suo ruolo e, inoltre (cosa ancora più importante), sulla necessità di avere interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza dei tratti più critici, sia nelle sedi ufficiali di Commissione che nelle numerose chiacchierate informali che caratterizzavano i minuti prima e dopo delle sedute, ha sempre manifestato l'esigenza di procedere per le parti che non avrebbero compromesso le soluzioni alternative bensì, rapidamente, avrebbero assicurato subito le popolazioni e i territori interessati. Recentemente, prima di una seduta in 8a Commissione, disse ad alta voce: «Avete sentito che intervento duro, ma anche bello ha svolto il senatore Cervellini in Aula?». Io, nel ringraziarlo, gli risposi: «Presidente, ma lei non era in Aula. Come può dire questo?». Mi rispose: «Ero in ufficio a lavorare, per predisporre gli atti e parlare con gli auditi che convochiamo convochiamo in Commissione, ma seguo sempre il dibattito dell'Aula. Rispetto e ascolto quello che viene detto dentro l'Aula». Ed era assolutamente vero, perché interveniva nel merito delle cose che avevo detto in quell'occasione. L'ho ricordato perché questo mette in luce una caratteristica di cui spesso discutevamo: quella di un rigore della politica che spesso non c'è più, dello studio e dell'ascolto che, anche nel confronto aspro, anzi tanto più, non deve venire meno. Oggi è raro trovare queste figure e non è assolutamente nostalgia canaglia quella che mi muove a svolgere queste considerazioni, niente affatto: è la necessità, tutta proiettata nel futuro, di ricostruire nel confronto anche duro, fatto di visioni e proposte nettamente alternative, il rispetto delle idee dell'avversario, della lealtà di fondo, figlia della profondità dell'essenza della conoscenza, non dell'improvvisazione e di una battuta più o meno indovinata. E sì che non gli mancava l'ironia. Anzi, ricordo innumerevoli punteggiature esilaranti e straordinarie per tempistica e profondità. Tempo addietro gli dissi, in una di queste chiacchierate in libertà: «Sai, Altero, nel 1984 ero molto giovane. Ero un giovane comunista. La morte di Enrico Berlinguer mi segnò profondamente così come, il giorno prima dei funerali, vedere in fila, come un comune cittadino e insieme a migliaia di compagni e compagne, Giorgio Almirante che andava ad onorare la figura dell'avversario nella camera ardente allestita in via delle Botteghe Oscure. Lo faceva lui, Almirante, il più netto dei suoi avversari. Oggi dobbiamo uscire dal maledetto pendolo della nostra attuale quotidianità che oscilla fra odio fazioso e inciucio spregiudicato». Ricevetti, perciò in quell'occasione, una lezione di vita e per questo, con assoluta modestia, senza voler fare alcun paragone diretto, porgo le più sentite e sincere condoglianze ai suoi cari, ai familiari, agli amici di vita e di partito, che hanno avuto la fortuna di poter ammirare e di essere accanto tanti anni ad Altero Matteoli. Lo faccio a nome mio personale e del Gruppo Sinistra Italiana-Liberi

Signora Presidente, colleghi, ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Altero Matteoli, un'uscita di scena resa più dolorosa per la maniera drammatica con cui è avvenuta: una vita spezzata, tanti progetti e iniziative lasciate sospese. Con lui senza dubbio viene meno uno dei grandi protagonisti della politica italiana degli ultimi venti anni e in particolare del centrodestra; di quel centrodestra, il cui ricordo porto nel cuore, nel quale varie tradizioni politiche erano riuscite a trovare una felice amalgama attorno alla figura di Silvio Berlusconi,

Altero Matteoli, anche se proveniva da una formazione culturale e politica diversa dalla mia, non l'ho mai sentito lontano e distante e, quando all'inizio di questa legislatura abbiamo intrapreso strade diverse, il suo comportamento è stato sempre improntato alla correttezza e al rispetto reciproco; questo perché era un uomo delle istituzioni, capace di fare politica senza urlare, ponendo sempre innanzi questioni di merito che non tracimassero o scadessero nel personale o nell'offesa.

Mi piace ricordare oggi proprio questo di lui, del suo essere politico, e mi spiace che non potrà essere un protagonista impegnato in questa difficile e delicata tornata elettorale: nel momento in cui il Paese rischia di scivolare lungo il piano inclinato del populismo, dell'esasperazione e della intolleranza, la sua saggezza, il suo realismo ma soprattutto il suo essere una persona perbene sarebbero state qualità preziose. Signora Presidente, sono profondamente cristiana e cattolica e so che Altero è già nel paradiso dei giusti. Da lì saprà ancora essere l'uomo delle istituzioni e sarà punto di riferimento per chiunque lo ha conosciuto e amato. Signora Presidente, mi lasci esternare alla famiglia e a tutto il Gruppo di Forza Italia del Senato il cordoglio di tutto il Gruppo di Alternativa Popolare.

Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Altero se ne è andato se ne è andato lasciandoci sgomenti, attoniti, increduli, lasciando un senso di profondo turbamento, ma anche di grande solitudine. Indipendentemente dai colori politici, le parole che ho ascoltato qui in Aula e che non sono frutto della circostanza, attesa l'autorevolezza di chi le ha pronunziate,

è frutto di una profonda convinzione della qualità che ha accompagnato questo nostro amico nel corso della sua storia politica e umana. Siamo stati tutti testimoni - io con tanti di voi in queste legislature - della qualità di Altero, nella sobrietà espressa in modo straordinario, una sobrietà nel linguaggio che era asciutto. Era un uomo che amava più ascoltare che parlare, dotato di un grande senso di equilibrio, di pacatezza, di competenza, di talento, ma anche di una profonda fede valoriale. Sono le doti che accompagnano un politico e ne fanno un uomo delle istituzioni che merita di essere ricordato. Ma dietro quello sguardo apparentemente severo o burbero - come ha detto l'amico Zanda - c'era di fatto la pacatezza del linguaggio e il suo volto si illuminava ogni qualvolta ci si intratteneva a parlare, dentro e fuori le Aule del Parlamento. Dopo Pinuccio Tatarella, credo che in effetti bene è stato definito come il «Ministro dell'armonia», perché con Altero non si poteva non andare d'accordo, perché era l'uomo dell'accordo. Era l'uomo che riconosceva riconosceva alla politica il valore del dialogo come condizione irrinunciabile per costruire un progetto oltre gli schieramenti, oltre le faziosità politiche; una prospettiva che consegnasse al Paese la qualità del lavoro che si svolge qui. Aveva detto più volte che, nella politica, il momento più bello è quando un avversario ti cerca per riconoscere il tuo valore. E ancora, aveva detto che in politica nessuno vince mai completamente e nessuno perde mai completamente, a significare che in politica devono sempre prevalere il buon senso e la strada della mediazione per trovare i punti Credo che questo sia il lascito di Altero che resta nel nostro cuore e nel nostro ricordo. Quelli che trattano di grandi cose testimoniano che «gloria dona al prode uomo una seconda vita», cioè a dire che, dopo la morte, la nominanza che rimane di buone opere mostra che si vive ancora dopo la morte. Queste parole, che il sommo poeta consegna sulla bocca di Brunetto Latini, mi inducono a dire che il modo migliore per onorare il nostro illustre collega e amico carissimo sta nella nostra capacità di conservarne il lascito e di trasformarlo in quotidiano esempio per restituire sempre di più dignità alla politica. Concludo rivolgendo alla famiglia il pensiero affettuoso di vicinanza e cordoglio del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ricordando quanto ho detto alla sua diletta moglie e ai figli: lascia a loro una grande eredità, ma lascia anche a noi un'eredità che si unisce all'orgoglio e al piacere di averlo conosciuto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con sentimento mi rivolgo alla famiglia, al Gruppo parlamentare e al partito di appartenenza per esprimere il cordoglio del Gruppo parlamentare Articolo 1-MDP-Liberi e Uguali. desidero associare al tributo politico e umano anche un mio personale cordoglio, che deriva da una frequentazione non proprio recentissima del senatore Matteoli. Ho conosciuto Matteoli tanti anni fa, entrambi nello svolgimento di funzioni istituzionali, e in quelle plurime occasioni ho avuto modo di constatare che, pur partendo da posizioni politiche molto distanti, il senatore Matteoli, il ministro Matteoli, non ha mai fatto mancare la capacità di esprimere lo spirito costituzionale della leale collaborazione. è sempre stata presente, anche quando chi vi parla e il ministro Matteoli erano portatori di opzioni programmatiche politiche divergenti. Già questo è un primo, importante riconoscimento a una figura umana e istituzionale. Il senatore Matteoli è stato un uomo delle istituzioni ma, per introdurre una riflessione politica alla quale assegno una qualche importanza, vorrei aggiungere che il senatore Matteoli è stato anche un uomo della Repubblica. La storia del secondo dopoguerra della destra italiana ci dice che, per un fase non breve della vita nazionale, la destra italiana ha agito nelle istituzioni, pur non riconoscendosi fino in fondo nella Costituzione e nella Repubblica. Poi c'è stata una fase importante, che è stata richiamata - e a me pare molto bello che quel richiamo sia stato fatto dal vice presidente Gasparri: c'è stata una fase nella quale la destra italiana, con la svolta di stringere un patto con la Nazione, volendo condividere in fondo i valori della Repubblica e della Costituzione. Quello fu un passo importante per la destra italiana, ma fu un passo importante per la Repubblica e fu un passo importante per tutti gli italiani; un passo che ha consentito di superare una - non l'unica - delle anomalie politiche italiane del secondo dopoguerra. Nel dire queste cose voglio rammentare anche che il senatore Altero Matteoli è stato protagonista di quella stagione e, proprio per il fatto di essere stato parte così rilevante in quella pagina della storia italiana, egli non è stato soltanto - come dicevo poc'anzi - un uomo delle istituzioni, ma è stato fino in fondo un uomo della Repubblica. Per questo suo contributo all'Italia e alla democrazia italiana credo che dobbiamo un grande riconoscimento democratico al senatore Matteoli. Con queste espressioni, che sono il frutto sicuramente di un riflessione politica, ma sono anche il portato di una mia personale esperienza umana, rinnovo

Signora Presidente, colleghi, voglio pronunciare solo qualche parola e mi scuso per la brevità del mio intervento, che non deve essere interpretata come mancanza di rispetto per la figura del collega,

e anche in quella occasione ho potuto apprezzare le sue capacità di dialogo con le autorità locali e con chi si stava occupando dell'opera. E il mio apprezzamento è aumentato anche in quella occasione.

avesse un buon rapporto personale, per quelle poche parole che si scambiano qualche volta al di fuori dei temi specifici della Commissione. Faccio le mie personali e sentite condoglianze alla famiglia per la perdita grave

il tuo amico Denis Verdini, ma la commozione, le lacrime, il dolore avrebbero sopraffatto le parole e, quindi, ha chiesto a me di farlo, ma il tuo amico è qui, dietro di me. Al mio fianco c'è un altro tuo grande e antico amico, che per molti anni ha condiviso con te una lunga militanza, ovvero Francesco Amoruso. Cari colleghi, la storia del ministro Matteoli è quella di una carriera politica di altissimo profilo e di lungo corso, in cui ha percorso la strada della destra italiana e del Movimento Sociale Italiano, dove ha ricoperto l'importante incarico di responsabile dell'organizzazione, poi con Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, vivendo la genesi del PdL e poi nel partito di Forza Italia, in cui è approdato. Era uno dei pochi politici veri che, al di là del colore politico, davvero piaceva a tutti.

Era veramente un uomo in mezzo alla gente, della gente e con la gente. Ha fatto il corso degli onori: è partito da consigliere comunale di un piccolo Comune, poi della grande Livorno per arrivare a fare il sindaco. Ha capito l'importanza del dialogo tra gli amministratori, i sindaci e i parlamentari. E poi ha ricoperto in maniera egregia e nobile, con grandi capacità unanimemente riconosciute, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente. Stiamo Stiamo ricordando un uomo che ha veramente portato le istituzioni ad altissimi livelli in ogni sua occasione. per questo che a nome mio, a nome del nostro presidente Denis Verdini, del suo amico Amoruso e di tutti i colleghi del Gruppo, abbracciamo la moglie Ginevra e i figli. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto, di essergli stati vicini e di averne condiviso molte battaglie. A voi il suo ricordo e il nostro abbraccio perché avete avuto la fortuna di averlo a fianco in tutti questi anni. Vi abbracciamo caldamente e calorosamente, perché riteniamo che in questo momento voi abbiate perduto veramente la cosa più preziosa e importante. CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei pensato e mai avrei voluto commemorare Altero Matteoli, un amico. un amico. Molti di noi, oggi, ricordano non solo un collega, ma soprattutto un caro amico. Personalmente ho conosciuto e ho apprezzato il suo lavoro nel non facile ruolo di Ministro, ruolo che ha svolto con grande competenza e capacità, riuscendo con abilità a circoscrivere le pressioni politiche, favorendo la reale necessità dell'opera e delle opere. Altero ha avuto il coraggio di promuovere e sostenere opere infrastrutturali attese nel nostro Paese da oltre trent'anni in quei territori che, per la loro marginalità, hanno sempre sofferto la fredda contrattazione politica. L'esempio di Altero è un insegnamento: la sua storia, la sua passione politica, la sua passione per il Governo. Alla fine, fare politica vuol dire sempre appassionarsi del Governo, dei problemi delle comunità, piccole o grandi che siano. non solo Ministro ma anche sindaco, che forse è il ruolo che più esalta le qualità di un uomo. Cari colleghi, in quest'Aula spesso la passione politica ci divide, la lotta a volte è aspra e priva di scrupoli; ma si creano anche rapporti di straordinaria intensità umana, basati su regole difficili da spiegare, favoriti della capacità di chi, come Altero, con autorevolezza e grande intelligenza riesce, appunto, a indirizzare la politica quotidiana su un terreno più nobile. A tale proposito, credo di poter affermare che, in questa legislatura in modo particolare, nel ruolo di Presidente della Commissione lavori pubblici, Altero sia riuscito a sorprenderci. Conciliare la sua importante funzione politica con quella di Presidente di Commissione non era semplice e per nulla scontato. Grazie alla sua saggia conduzione, ci ha messi in condizione di dare il meglio di noi stessi, maggioranza e opposizione. Grazie soprattutto a lui, abbiamo fatto, cari colleghi dell'8a Commissione, un buon lavoro. Siamo riusciti ad armonizzare le differenze, favorendo il buon senso nelle scelte. La sua riconferma alla Presidenza di questa Commissione parla da sé. In questo momento in cui l'antipolitica è sempre più forte e tutto sembra accanirsi contro di noi, l'esempio di Altero, ancora di più in questa legislatura, cari colleghi, ci insegna che, se vogliamo riconciliarci con il Paese, la strada è questa. Non c'è nulla di nuovo da inventare, se non riscoprire il servizio alla comunità e l'umiltà del contatto con la gente e la ricerca della concordanza, proprio come Altero ha perseguito nella sua lunga carriera politica. Cari colleghi, signora Presidente, a nome della Lega Nord voglio esprimere la nostra vicinanza ai familiari in questo momento di grande tristezza, sperando che il tempo possa in parte colmare il vuoto che Altero ci ha lasciato.

sono qui oggi per un compito al quale mai avrei voluto adempiere e che mai avrei pensato di dover assolvere. Lo dico innanzitutto ai famigliari, ai collaboratori di Altero, al Gruppo di Forza Italia, ai quali vanno le mie personali condoglianze e quelle del Gruppo della Federazione della Libertà. In circostanze come questa si rischia sempre un po' di scivolare nella retorica, e so perfettamente di correre questo pericolo nel dire che se alcuni di noi hanno perso un amico fraterno, tutti abbiamo perso un collega stimato e benvoluto, le istituzioni della Repubblica hanno perso un servitore di valore e la politica ha perso un interprete appassionato e leale. Soprattutto, non credo che sia un esercizio di mera apologetica affermare che la figura di Altero ha incarnato la politica nel suo significato più nobile. La sua vicenda biografica ha attraversato le generazioni e le epoche; ha seguito le evoluzioni del quadro politico fin dai tempi del Movimento Sociale, senza mai smarrire il senso della militanza come cifra di un impegno; ha sdoganato molto più di altre biografie, che pure hanno avuto opportunità ancora maggiori, quei fattori di rettitudine, *gentilhommerie,* conciliante rigore che erano propri della sua cultura di origine e che sarebbe il momento che tutti nel Paese, anche coloro che ne sono fieri avversari ideologici, riconoscessero. Altero è caduto da militante, su quella strada maledetta che aveva battuto mille volte e che, dopo un periodo di ingiuste amarezze, lunedì era felice di tornare a percorrere per lanciarsi in una nuova campagna elettorale. E da militante ha vissuto i tanti ruoli che la vita lo ha portato a ricoprire, dall'era del Movimento Sociale all'avvento del centrodestra di governo che lo ha visto indiscusso protagonista, fino a questa tormentata legislatura che ancora una volta lui ha attraversato con il suo tratto al tempo stesso identitario e mediatore. Il punto è che Altero amava la politica; la viveva con istintuale passione ma ne conosceva le regole e le sapeva rispettare. Per questo godeva del rispetto di tutti, amici e avversari, al punto - è stato detto - di essere riconfermato Presidente di un'importante Commissione del Senato pur essendo un esponente dell'opposizione. Sempre per questo, nei momenti più difficili per la nostra parte politica, scendeva in campo con la sua attitudine alla composizione delle controversie senza cedimenti sul piano ideale, aiutato in ciò da una carica umana di rara intensità. In questa legislatura lo si ricorda ad esempio impegnato con gli amici Paolo Romani e Maurizio Gasparri a cercare di evitare in ogni modo la dolorosa separazione in seno a quel Popolo della Libertà che considerava, a mio avviso a ragione, una delle più felici intuizioni politiche del nostro tempo. E più di recente, quando la diaspora sembrava irreversibile e il centrodestra avviato a una inesorabile deflagrazione, era lì a coltivare un sogno unitario, considerato allora un esercizio di non lucida follia;

Ho avuto la fortuna di esserne testimone diretto, perché nelle iniziative pubbliche messe in campo per agevolare questo percorso Altero mi ha dato l'onore di essere al suo fianco, consentendo alla mia fondazione di collaborare con la sua, che era per lui motivo di grande orgoglio, stimolo di pensiero politico e fucina di calore umano, e che saprà andare avanti in suo nome. Altero ci mancherà, tanto. Ci mancheranno la sua passione, la sua saggezza la sua autorevolezza. Ci mancherà l'irrefrenabile ironia con cui sapeva condire anche i passaggi più duri e che, per lui che aveva un profondo rispetto degli avversari in politica, diventava prorompente quando si trattava di infierire sugli avversari nel campo del calcio. Lui juventino fino al midollo, io tifoso accanito del Napoli, eravamo soliti sfotterci a vicenda a ogni giornata di campionato. In occasione dell'ultimo rovescio inflitto dalla sua Juventus al mio Napoli, egli ha avuto invece pietà. Si è astenuto dallo sfottere, e il giorno dopo mi ha chiesto se avessi apprezzato il gesto. Ovviamente ho capito che era solo un modo diverso di sfottere; un modo lieve e affettuoso, come Altero sapeva essere in politica e nella vita e come lo ricorderemo per ogni giorno a venire. Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, non ho avuto con Altero Matteoli quella familiarità e quella consuetudine che consentono il ricorso a un termine così impegnativo come amico. Tuttavia, ho chiesto di parlare per ricordare in questa sede due episodi della nostra pur esile relazione, che ritengo essere non semplicemente due dettagli, bensì fatti rivelatori di elementi significativi e profondi della sua personalità. Il primo appartiene alla cronaca politica nazionale di questo Paese e risale al 2006, quando, nel mese di luglio, il Parlamento approvò una legge controversa e, tuttavia - a mio avviso - così importante e sacrosanta come il provvedimento di indulto. Altero Matteoli fu l'unico - sottolineo l'unico che votò a favore del provvedimento e che, solitario e fiero, ne rivendicò la saggezza nei mesi e anni seguenti. E fu tra i pochissimi

Quell'episodio - a mio avviso - è significativo di una concezione delle libertà individuali e di una attenzione per i diritti della persona che non sono così diffusi all'interno del suo stesso schieramento. Il secondo episodio è più recente. Ritornato in Parlamento dopo molti anni, in questa legislatura venni da lui interpellato per avermi sentito attraverso Radio Radicale, una sorta di elogio della militanza. Ci incontrammo a pranzo ed egli mi parlò, con grande intensità, della sua concezione della politica. E, con un atteggiamento fatto anche di una certa audacia nel superare d'uno balzo solo antichi confini e perimetri, parlò di quella generazione - così la definiva - fatta di coloro che avevano attaccato i manifesti sui muri, e cioè di coloro che avevano interpretato la militanza come una sorta di relazione stretta tra vita privata ed esistenza pubblica. E con ciò rivelava una sorta di solidarietà con quanti, non solo diversi da lui per posizioni culturali e politiche, ma spesso a lui a lui contrapposti - e negli anni precedenti, in anni ormai lontani, la contrapposizione non era solo drastica e radicale, ma spesso, com'è noto, era contrapposizione aggressiva - rivelavano, ai questa sorta di comunanza nella medesima idea della politica come pienezza dell'agire umano, e cioè come passione, termine che ricorreva nelle sue parole, pur abitualmente così sobrie, addirittura asciutte e spesso intenzionalmente e volutamente disadorne e disincantate. In quella conversazione (che ricordo con precisione, anche se sono passati ormai alcuni anni) volle, appunto, illustrarmi questa idea della militanza che sapeva

un istinto, una relazione stretta tra vita privata e vita pubblica, dedizione e sacrificio: la politica come qualcosa di terribilmente serio. Bene: questa concezione della militanza, in un tempo che vede la politica così denigrata, così frammentata, così mortificata, penso che resti un'importantissima lezione, che vale per tutti noi, al di là di ogni schieramento, al di là di ogni contrapposizione, al di là di ogni divergenza. Penso che di questo tutti possiamo essergli grati.

commemorato doverosamente l'amico Altero. Non potevo, però, sottrarmi, anche per mia storia personale, dal rassegnare qualche mia riflessione e ricordo nei confronti dell'amico; un amico che considerava la politica una politica dei valori solidi: lo spirito dell'abnegazione, del confronto, del rispetto. un politico di alta scuola, che mi ha visto al suo fianco, nella XV legislatura, da Presidente del mio Gruppo (lui Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, seduto in questi banchi), in un'azione di contrasto politico, a volte acceso, ma sempre corretto, nei confronti di un Governo politicamente debole per i numeri parlamentari.

confronto e della responsabilità, trovare punti di sintesi, in una logica di convergenze, per fare emergere le contraddizioni di un'azione di Governo che lamentava una propria eterogeneità di forze politiche. Con Altero ci siamo confrontati spesso, da lui ho appreso la logica della riflessione e, a volte, anche della comprensione nei momenti di forte dialettica politica parlamentare.

dell'amore nei confronti della propria gente. È caduto sul campo, come ha detto l'amico Maurizio Gasparri, lavorando per il territorio, guidando la sua autovettura, mentre girava la sua terra. Si sarebbe incontrato con i suoi militanti,

della capacità di riflessione e del rispetto nei confronti dell'avversario. Altero era un uomo di destra, ma la destra non significa necessariamente estremismo: affatto. È una destra di valori, per la quale si è parlato del dopo Fiuggi, da parte del collega Manconi e altri;

Quante volte ho assistito a riunioni ristrette del mio partito in cui la parola di Altero Matteoli era quella del saggio, dell'uomo ascoltato dal *premier* Silvio Berlusconi, della

Esprimo ancora una volta alla famiglia il saluto e l'abbraccio del Senato. *(Applausi).* Si conclude qui la commemorazione del senatore Altero Matteoli.

il provvedimento che stiamo esaminando è nato da una riflessione molto condivisibile. Si parla spesso del fenomeno delle donne che vengono uccise dai loro mariti, compagni, *ex* mariti ed *ex* compagni, creando non soltanto una evidente tragedia in sé per la donna che viene uccisa, ma lasciando anche degli orfani in condizioni particolarmente difficili, hanno perso la madre in un modo e il padre in un altro. Di conseguenza, si è deciso di istituire delle misure, tutte condivisibili, per i bambini che si trovano in questa situazione. situazione. L'esigenza che ho descritto ha la sua piena giustificazione. Quante volte una legge, del tutto giusta e del tutto doverosa, è partita anche solo per un singolo caso che ha evidenziato qualche carenza nella legislazione o, comunque, l'esigenza di rinnovarla, di introdurre nuovi provvedimenti o di cancellarne di vecchi? Però il provvedimento, anche se nasce in questo modo, deve essere poi studiato in modo che abbia il suo equilibrio, il suo senso, i suoi criteri di costituzionalità, e

che si trovano ad aver perso, come ho detto, la madre in un modo e il padre in un altro; la madre purtroppo per sempre mentre il padre non sempre

costui va giustamente in carcere, anche a lungo, e spesso gli viene tolta la potestà genitoriale, per cui questi bambini si trovano in una situazione particolare. Tuttavia, non possiamo ritenere non possiamo ritenere meno meritevoli di tutela tutti i bambini che vengono a trovarsi, a seguito di reati di reati violenti, in una situazione analoga, improvvisamente, con la possibilità non infrequente, né per quanto riguarda il cosiddetto femminicidio né per quanto riguarda altri tipi di reati violenti, che possano anche aver subìto essi stessi direttamente un trauma, quindi non solo la perdita del genitore o dei genitori, ma anche traumi per essere stati forse o avere percepito in modo comunque diretto lo *shock* di questo atto violento. Le nostre richieste sono state molto semplici. C'è chi addirittura chi ha parlato di ostruzionismo. No, noi abbiamo semplicemente difeso un criterio che ci sembra incontrovertibile e cioè che, se si dà una particolare tutela ai bambini che hanno perso i genitori in questo modo, bisogna dare la tutela a tutti gli orfani che sono stati privati dei genitori a seguito di reato violento. Al momento in cui un bambino perde il padre e la madre, che l'uccisore sia stato l'ex *partner* della madre o un rapinatore o un terrorista, davvero non riusciamo a percepirne la differenza, ed è davvero difficile sostenerla.

gruppo di bambini, è che si voglia fare una norma che va dietro alla cronaca. Noi sappiamo che molti fenomeni, in particolare di crimine,

frequenza con la quale ne viene data notizia con grande rilievo dai mezzi di informazione. Noi sappiamo che qualunque omicidio è un fatto gravissimo, particolarmente esecrabile; è particolarmente esecrabile quello di una donna,

sostenitori, iniziatori di norme che diano adeguato sostegno e prendano le misure opportune per proteggere i bambini che si sono trovati privati dei genitori a causa di femminicidio di donne che vengono uccise dal *partner* o dall'ex *partner*. Non possiamo però per questo chiudere gli occhi; anzi deve essere l'occasione per prenderci cura anche di situazioni che hanno una conseguenza del tutto uguale,

a seguito di crimini violenti, ma che non rientrano negli stretti parametri previsti dalla norma che stiamo discutendo, debbano fare ricorso alla Corte costituzionale, la quale dovrà affermare ciò che è assolutamente ovvio, cioè che non si può fare differenza tra il soggetto che ha ucciso la madre di una persona, per stabilire se quest'orfano è meritevole di attenzione da parte della legge. non deve affermarlo la Corte costituzionale, lo capiamo facilmente noi, basta avere la buona volontà. Noi siamo per fare tutto il possibile perché ciò venga fatto. C'è lo spazio per approvare il provvedimento anche alla Camera, certo che però bisogna farlo. Bisogna volerlo, altrimenti approviamo una legge monca, per un atto di giustizia diventa un atto di ingiustizia nei confronti dei bambini che si trovano nelle stesse situazioni, sia pur non con i parametri che in quel momento sono stati decisi.

alla ragione di fondo, alla *ratio* di questo provvedimento, sottolineando il fatto che sul tema della violenza alle donne e ai minori chiudiamo la legislatura

in quanto viola il principio di uguaglianza. È un cambio di passo culturale e giuridico. Il nostro Parlamento è stato tra i primi tra i primi in Europa a ratificare la Convenzione. Ricordo l'emozione di averlo fatto qui in Senato, per conto della Commissione esteri in quel mese

per i centri antiviolenza e, da ultimo, la stessa Commissione sul femminicidio. Stiamo compiendo uno sforzo congiunto per istituire una cabina di regia, al fine di coordinare prevenzione e sostegno, dalla scuola di polizia, al pronto soccorso, al controllo della pubblicità. Dicevo che l'Italia - mi interessa questa dimensione internazionale che spesso non valorizziamo abbastanza - è il primo Paese in Europa ad affrontare con questa ampiezza e natura la questione.

a specificarlo meglio. Parlo cioè di quelle relazioni intime che non sono solo legate alla consanguineità, ma a un'idea profonda di relazionalità affettiva che, per definizione, richiede e chiama affidamento, fiducia, rispetto e protezione, cioè tutto quello che

d'onore. Lo spirito e la ragione che ci muovono sono infatti quelli di archiviare quella cultura del delitto d'onore che cancellammo tardivamente nel 1981, ma che riemerge con odiosa forza, in qualche modo subliminale, quando si afferma da tutte le parti,

Per terminare vorrei ricordare il nostro contributo internazionale, di cui abbiamo potuto verificare l'efficacia quando abbiamo partecipato con la collega Puglisi e la collega Fabrizia Giuliani al dibattito voluto dal Parlamento europeo su questo tema. Vi dico solo questo: stiamo tornate sconfortate da Bruxelles per le resistenze dei Paesi dell'Est, in *primis* della Polonia, a ratificare la Convenzione.

se si rafforzano le relazioni affettive basate sulla libertà e la dignità. Quindi concludo dicendo che dobbiamo fare attenzione anche a queste radici quando parliamo del pericolo del populismo europeo

Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve anche alla luce del fatto che è importante che il nostro Parlamento completi, nel corso di questa legislatura,

e andiamo ulteriormente a rafforzare quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione di Istanbul e, insieme, andiamo ad avvalorare e rendere legislativamente concreta

la quantità dei soggetti minori che devono essere tutelati dallo Stato. Ricordo infatti al Senato che proprio uno degli emendamenti, a prima firma della collega Puglisi,

Tale Fondo è disponibile per le vittime, in particolari minori, dei reati mafiosi, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti, esso si inserisce, grazie a questo emendamento, un'ulteriore e importantissima categoria, che ha visto negli ultimi quindici anni 1.628 bambini o ragazzi,

agli orfani di crimini domestici e di femminicidio, ovvero a 1.628 bambini o ragazzi nel corso degli ultimi quindici anni. Ho voluto fare questo intervento, perché ho seguito l'*iter* di questo disegno di legge molto importante,

di fronte ai tre figli, bambini e ragazzi, tra cui la più grande, Nancy, che da allora si mantiene con una borsa di studio e ha deciso, invece di procedere come immaginava di poter fare, con una

perché molto spesso non si è riusciti a prevenire e ad intervenire in tempo ed ecco perché ce ne occupiamo anche con un fondo ulteriore e con una volontà di inserimento di un progetto legislativo. Voglio farlo, poi, per Stefania Mattioli, la mamma di Claudia Ferrari,

Da due anni a questa parte le sta accudendo come una madre, da sola, rinunciando a una parte fondamentale del proprio reddito, perché doveva lavorare e così facendo ha dovuto, almeno almeno parzialmente, interrompere la propria attività lavorativa. Dunque questo Fondo, insieme con questo disegno di legge, dovrebbero andare finalmente a lenire le sofferenze gravi, anche di tipo economico, che hanno subìto, purtroppo, ancora a maggior danno di quanto già subìto psicologicamente, questi orfani di femminicidio. Voglio ringraziare particolarmente coloro che hanno contribuito alla stesura di questo disegno di legge che contiene due aspetti che rappresentano un cambio di paradigma che io credo

per il padre o comunque il soggetto che si è reso responsabile del femminicidio, oggi prevede una maggiore tutela per il semplice fatto che abbiamo inserito immediatamente applicabile - quindi ancora prima della prima sentenza di primo grado - il fatto che vi sia una sospensione degli aspetti successori a favore dei figli minori che vanno tutelati e vanno difesi da padri che spesso vanno difesi da padri che spesso fanno persino atti privati presso notai e avvocati per togliere ai propri figli le possibilità di successione rispetto alla pensione della madre o alle proprietà immobiliari della famiglia.

con un'innovazione dal punto di vista del procedimento penale, nel nostro codice penale si inserisce un meccanismo che obbliga i

perché questa è l'obiezione che ci è stata posta in Commissione e molto probabilmente ci verrà detto, ove mai dovessimo essere particolarmente incidenti nella discussione, che, sì, è vero, ci sono degli errori ma intanto variamo questa legge e che agli errori si porrà rimedio successivamente. Quello che ci è stato detto tante e tante volte in quest'Aula, ogni qual volta abbiamo varato una legge costretti dai tempi.

a tutti i minori il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore, ovvero dalla persona con cui il genitore minore stesso convive sicché, in ragione di questo fatto omicidiario, il minore viene a perdere completamente il suo ambiente familiare - l'ha detto la relatrice e l'ha detto da ultimo la senatrice Puppato - noi non avremmo avuto alcuna obiezione al varo di questo disegno Il problema di fondo è che esso dice cosa molto diversa e siccome nell'ascoltare, sia qui in Aula che fuori, qualche intervento o qualche notazione,

e si apprestino a dare il proprio voto basandosi sulla suggestione giornalistica o propagandistica politica, utilizzerò quel poco di tempo che ho a disposizione per cercare di spiegare bene il concetto. L'articolo 1 di questo disegno di legge afferma che viene dato il gratuito patrocinio in deroga rispetto alla disciplina vigente al minore il cui genitore - e qui vi pregherei di voler prestare un po' di attenzione - viene ucciso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato,

Abbiamo provato a dire, in Commissione, che c'è una lacuna di non poco conto e cioè quella relativa al genitore che non è coniuge e che non è convivente, ben potendosi verificare il caso di un genitore che non abbia sposato l'altra parte o non abbia convissuto con l'altra parte, quindi il minore il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore non coniuge e non convivente non potrebbe godere dei benefici - corretti e giusti - di questo disegno di legge. La seconda obiezione che abbiamo fatto in Commissione

in maniera del tutto sganciato, da un rapporto di convivenza che l'assassino ha con il minore. Farò degli esempi, così siamo tutti più contenti.

Quell'assassino non ha mai avuto alcun rapporto con mio figlio, il quale vive tranquillamente con sua madre; in altri termini il genitore di quel bambino (cioè io)

«dal convivente o dal *partner* dell'unione civile che abbia avuto convivenza con il minore». Se però il minore non ha mai avuto alcuna forma di convivenza o di contatto con l'assassino del genitore, mi spiegate la ragione di questa tutela, dal momento che l'ambiente famigliare, a cui qualcuno ha fatto riferimento, sostanzialmente non si è rotto nella sua completezza?

all'articolo 3 e all'articolo 4 è previsto che il pubblico ministero possa sequestrare i beni dell'assassino a tutela delle pretese risarcitorie del minore

Abbiamo chiesto, siccome questa norma non costa nulla, che almeno queste due norme venissero estese a tutti i minori il cui genitore o i cui genitori vengono meno a seguito di un fatto delittuoso. Mi volete voi spiegare la ragione per la quale il pubblico ministero è obbligato a sequestrare i beni nei casi di cui all'articolo 1 e invece può non sequestrarli nel caso in cui i genitori siano morti per un qualsiasi altro fatto delittuoso? Quel minore, i cui genitori sono morti al di fuori di un contesto familiare, non costando nulla la norma, ha o no diritto ad avere un minimo di tutela simile a quella degli altri minori? Stiamo creando, per problemi propagandistici e bandieristici, un'incredibile disparità di trattamento tra i minori? E quando questa posizione verrà prospettata all'interno di un procedimento penale, non pensate voi che a qualcuno potrà venire in testa di sollevare - correttamente, a mio avviso - un'eccezione di illegittimità costituzionale?

noi auspichiamo che si possa ragionare, in quanto alcuni emendamenti sistemerebbero e completerebbero il quadro. È chiaro che apporre emendamenti adesso, in seconda lettura, in questo momento della legislatura,

di modificare, di rendere più completa e definitiva questa proposta di legge, tanto, se dobbiamo ritrovarci il 27 o il 28 dicembre, comunque prima di Capodanno, la Camera potrà rimodellare e ridefinire questo provvedimento e noi definiremo, invece, la manovra di bilancio.

mettendo sulla bilancia, da una parte e dall'altra, ciò che c'è di positivo e ciò che ancora manca o che c'è di negativo, la bilancia ci sembra che penda dalla parte

reati consumati all'interno della famiglia e, il più delle volte, all'interno della stessa coppia. Non c'è dubbio che questo tipo di reato crea un problema indissolubile legato agli orfani, che il provvedimento che stiamo esaminando dovrebbe tentare di tutelare maggiormente. Spesso sono minori, si trovano senza madre e, nel caso dell'omicidio domestico, con un padre in carcere, per cui sono le vere vittime: si definiscono vittime secondarie, ma sono le vere vittime di questo tipo di reato. necessario un provvedimento che andasse in questa direzione, che tutelasse proprio questo tipo di orfani.

potrebbe anche pagare tranquillamente delle spese. Pertanto, non si è definita tutta la casistica; capisco che la casistica è infinita, ma si poteva aggiungere qualche «salvo il caso in cui» il minore abbia ancora un genitore vivo, in grado di supportare, per questioni di capacità reddituale, i costi di un processo.

Qualora il reato sia commesso dal coniuge, contro l'altro coniuge, ancorché separato legalmente, da una delle parti civili o dalla persona legata da relazione stabile o affettiva, ovvero il compagno convivente. Dal punto di vista processuale, la proposta intende dare maggiore tutela ai figli delle vittime di questi reati. Diciamo che si prevede innanzitutto un diritto al risarcimento del danno, si rafforza, in questo caso, la tutela dei figli e si stabilisce che il pubblico ministero avrà l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni, anche nel caso in cui l'indagato sia tale e il processo non sia definito, in ogni stato e grado. Viene modificato l'istituto della provvisionale, nel senso che

La proposta interviene su un altro istituto, quello dell'indegnità a succedere, che è stato ben puntualizzato dal collega Palma.

sarebbe un paradosso, pertanto è giusto dire e scrivere - *ad abundantiam*, in questo caso - che è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato. Si eviterebbe così che gli altri eredi dovessero promuovere un'azione civile per arrivare a questo risultato.

privilegi sono i figli di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio, come i grandi invalidi per cause di guerra. Bene: anche i figli

che il marito che ha ucciso la moglie possa poi beneficiare anche dei diritti di lei, che non c'è più. Alle Regioni e alle autonomie viene demandato il compito di promuovere servizi informativi e assistenziali. vengono garantiti il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro e si prevede anche un'assistenza medico-psicologica per tutto il periodo che serve per il pieno recupero del loro equilibrio psicologico. È corretto parlare

in caso di violenza domestica: si parla di incesto, maltrattamenti ai familiari, infanticidio, lesioni personali e via dicendo. E infatti, alla fine si prevede anche che gli orfani avranno la facoltà di richiedere la modifica del proprio cognome, nel caso in cui coincida con quello del genitore che viene condannato in via

vittime del reato e si va nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Speriamo prevalga il buon senso e che si superino steccati politici.

Signor Presidente, il 18 dicembre scorso a Parabiago, in provincia di Milano, Simona Forelli, una donna di trentatre anni, è stata uccisa a coltellate dal proprio compagno davanti ai suoi due figli, rispettivamente di diciassette Si tratta della ottantesima donna vittima di femminicidio che ricordiamo in quest'Aula a conclusione di una staffetta durata un anno e mezzo, che io ho promosso e alla quale hanno partecipato una cinquantina di altre senatrici e senatori, che ringrazio. Ricordando queste donne tante volte abbiamo visto che lasciavano dei figli, e ci siamo preoccupati del loro vissuto e della loro situazione dopo l'uccisione violenta della madre. Di questo tema comincia, meritoriamente, ad occuparsi questo disegno di legge. Le donne che subiscono violenza dal proprio *partner* spesso temono per la sicurezza dei loro figli, durante la relazione e anche dopo la separazione, quando non sono più presenti a mediare per loro. È la paura per il destino dei figli che rende ancora più angosciosa e difficile la loro situazione. Le loro paure non sono infondate. La ricerca, anche accademica, ha da tempo mostrato che i padri che usano violenza sulle madri dei loro figli tendono ad utilizzare l'abuso e altre tecniche di controllo anche nei confronti dei bambini. Con riferimento agli studi effettuati negli Stati Uniti, in media, entrambe le forme di violenza sulla donna e sui figli sono state riscontrate nel 40 per cento delle famiglie studiate. Anche la probabilità di essere vittime di incesto è risultata 6,5 volte maggiore per le figlie degli uomini maltrattanti. Ma non è necessario che vi sia violenza diretta, fisica o sessuale, sui bimbi, perché questi riportino un danno dalla esposizione alla violenza domestica. I bambini vittime della cosiddetta violenza assistita possono mostrare problemi, emotivi e comportamentali, analoghi a quelli dei bambini vittime di violenza diretta. Per questo è molto importante che l'articolo 9 del disegno di legge che stiamo esaminando rechi disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica per tutto il periodo necessario per il pieno riequilibrio psicologico degli orfani di femminicidio. Così come è stato importante che il reato di violenza domestica, introdotto con il decreto-legge n. 93 del 2013, veda come circostanza aggravante il fatto che la violenza sia esercitata in presenza o in danno di un minore. La violenza assistita è aumentata nel nostro Paese. La percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre, secondo l'indagine dell'Istat, è passata da 60,3 del 2006 ha 65,2 per cento Vi è poi un'importante e noto fenomeno: la trasmissione intergenerazionale della violenza. Sempre secondo l'Istat, il figlio che ha assistito alla violenza tra i genitori il figlio che ha assistito alla violenza tra i genitori diventa autore di violenza a sua volta nel 22 per cento dei casi e lo diventa nel 35,9 per cento dei casi se ha subito lui stesso, da piccolo, violenza fisica. Oggi parliamo di riparazione dei danni subiti dagli orfani di femminicidio, ma ancora più importante è la prevenzione che dobbiamo mettere in atto. Dobbiamo combattere perché le donne che temono per i propri figli siano credute e non succedano più fatti come il figlicidio di cui è stato vittima Federico Barakat, ucciso a 8 anni nel 2009 dal padre nelle stanze dei servizi sociali a San Donato Milanese, durante un incontro protetto. La madre aveva chiesto disperatamente la sospensione di quegli incontri che esponevano il figlio a un grave pericolo, ma le si era risposto con la minaccia di allontanare il figlio anche da lei, accusata di voler ledere la figura genitoriale paterna, la cui difesa è stata quindi anteposta alla difesa della stessa vita di Federico. Il caso è ora all'attenzione della Corte di giustizia europea, in un ricorso reso procedibile nel novembre scorso, in cui il Governo dovrà rispondere su indagini chiuse forse troppo frettolosamente, su errori di valutazione, sul risarcimento da riconoscere. Ma ancora più importante, in un'ottica di prevenzione, è mettere in conto misure non solo di formazione degli operatori, ma anche di revisione normativa, in particolare evitando il ricorso all'adozione condivisa in tutti i casi in cui un genitore - sappiamo che si tratta generalmente del padre - si sia reso responsabile di violenza nei confronti dell'altro genitore. E questo è già programma per la prossima legislatura.

spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclamava e attendeva da parecchio tempo. scritto del mio intervento, ma voglio ricordare le tante novità positive, che già tanti hanno menzionato in Aula. Penso innanzitutto all'introduzione del gratuito patrocinio; penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il colpevole di uxoricidio; penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado. Come anticipato all'inizio del mio intervento è con grande soddisfazione che plaudo ai lavori del Parlamento per aver deciso di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, al fine di sostenere queste giovani vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure di sostegno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita dal trauma che si trovano costretti ad affrontare. Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati. Come preannunciato, chiedo

per ragionare insieme a voi su che cosa fare. La senatrice mi ha chiesto qualche giorno fa, in una intervista radiofonica, come avrei votato (perché questo è il vostro modo di ragionare). Glielo dico ora: forse a favore; forse non partecipo; forse voto contro. Perché? A favore, in quanto certamente ci sono alcune situazioni che vengono disciplinate; ci sono errori, perciò dovrei votare contro; ci sono possibilità di correzione, perciò potrei astenermi. Quando abbiamo votato la legge sulla violenza sulle donne, tutti i Gruppi hanno riconosciuto tre errori in

sui testimoni di giustizia: non ho presentato emendamenti e l'ho sostenuta fino in fondo, perché questo è il modo di fare politica. Allora, verifichiamo che cos'è che non va in questa legge. Abbiamo cambiato qualcosa con i nostri emendamenti? Abbiamo tolto qualcosa ai minori che si volevano tutelare? No, con i nostri emendamenti venivano tutelati questi minori e anche gli altri. Quali altri?

in questo caso, il figlio ha diritto, in base a questa legge, al gratuito patrocinio. E perché, se Tizia è un'estranea per lui? Allora, per quale motivo gli altri orfani, vittime di estranei, non devono avere la stessa tutela? È ridicolo l'articolo 1, con una copertura di 10.000 euro per il gratuito patrocinio. Sapete tutti che non è così:

sa che ci sono anche uomini ammazzati dalla compagna, dal marito di lei e così via. Questa prima norma, così come l'avevamo scritta con l'emendamento, cioè aumentando la dotazione,

all'articolo 5, quando si parla dell'indegnità a succedere, si afferma che la persona che ha ammazzato è sospesa della successione e siamo tutti d'accordo;

Questo è il curatore dell'eredità giacente. Avete capito questo cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini non avranno la disponibilità dei loro beni per tutto il tempo del processo penale. Abbiamo presentato un emendamento che correggeva questa ipotesi e dava la possibilità di nominare un curatore all'eredità giacente solo per la parte dell'assassino, perché attualmente la giurisprudenza e la dottrina non consentono di tener conto di una separata parte dell'eredità ai fini della curatela. Il punto è il seguente: volete mantenere ferme le altre questioni? Fate quello che volete, ma intervenite almeno su questo per salvare i minori. Mi rendo conto che non c'è tempo,

e voi volete bloccarli finché non ci sarà il processo penale. Siano bloccati solo i beni dell'assassino! Mi rendo conto che non abbiamo tempo, ma allora vorrei una risposta. Vorrei sapere: c'è un impegno, sperando che nella prossima legislatura, che anche se non ci fossimo noi, chiunque sarà presente in quest'Aula avrà la sensibilità di porsi il problema?

è la prima questione. La seconda questione è quella dell'eredità giacente: tutto il resto sono conseguenze, Non c'è nessuna opposizione al disegno di legge approvato alla Camera, si trattava di migliorarlo e di renderlo coerente con le norme e con l'ordinamento per garantire parità di diritti. Abbiamo Abbiamo tentato di spiegarlo in tutte le salse. Addirittura, la relatrice nel corso dell'esame in Commissione aveva detto che era d'accordo; poi, semplicemente perché, nella forma, come ho detto prima, non si potevano mantenere le due cose, ha detto che volevamo togliere le unioni civili. Ma che importanza ha?

nella nuova legge di bilancio, che ci arriverà domani o dopodomani, sarà necessario - mi insegnate - fare una correzione dell'articolo 1, che destina soltanto 10.000 euro. euro. Occorrerà fare una correzione. A questo punto, non sarà nemmeno possibile fare la correzione al bilancio, se non è stata fatta specificamente sul disegno

Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato in modo appassionato a questo utile dibattito. Sappiamo che i tempi sono tiranni su questo provvedimento, ma nel corso dell'esame degli emendamenti sono pronta a

Presidente, a questo punto ho un ulteriore problema: la relatrice si è resa conto del problema e ha detto che è d'accordo a esprimere parere favorevole sui miei ordini del giorno, che formalizzo. Credo che anche la senatrice Lo

è un disegno di legge che discrimina gli orfani, è punitivo nei confronti di tutta una serie di bambini che si trovano senza genitori ed è tale per una ragione ideologica.

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata» e qui il femminicidio non c'entra nulla, se permettete «o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza»

e un'offesa, perché i soggetti di questa legge avrebbero dovuto essere gli orfani. Anche nel caso di un omicidio stradale, se rimangono due bambini piccoli che perdono il padre e la madre, essi dovrebbero avere assistenza, perché sono rimasti orfani a causa di un reato, che abbiamo qualificato come omicidio. Il soggetto di Il soggetto di questa legge, però, non sono gli orfani, ma l'idea ideologica che una certa categoria di persone, che ha dei figli, possa avere più diritti degli altri. dal senatore Palma, che se una persona ha avuto un rapporto di *coniugio* venti o trenta anni prima e poi, per una serie di ragioni, arriva ad uccidere uno dei coniugi - fra le altre cose avendo egli stesso dei figli,

«I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore (...)». È quello che tutti avete detto e siamo tutti d'accordo: se un padre uccide la madre e il bambino si trova senza madre, con il padre in carcere, è certo che ha bisogno di tutta l'assistenza possibile e immaginabile.

Presidente, intendo illustrare gli emendamenti. Vorrei chiarire un concetto:

e cioè, sostanzialmente, minori il cui genitore viene ucciso dal convivente, ex convivente o quant'altro. Cosa contestiamo con gli emendamenti? Taluni errori tecnici. tecnici. Contestiamo principalmente un metodo, signor Presidente, perché quando ciò si poteva fare, cioè tre mesi fa, ci è stato detto che il testo sarebbe stato varato esattamente così com'è,

taluni sospetti di incostituzionalità che questo testo, a nostro modesto avviso, presenta. Comunque sia, Presidente, si vedrà poi in dichiarazione di voto. Una cosa però va detta: questo testo è sbagliato ed è dannoso per il minore con riferimento proprio all'articolo 5, relativo al tema dell'indegnità a succedere. Ve l'ha spiegato il senatore Caliendo. Con questo testo, l'eredità verrà bloccata e sostanzialmente, in ragione di tale blocco, verranno meno i beni beni a sostegno del minore. Noi volevamo dire solo questo, ma poiché dall'altra parte continuiamo a registrare il silenzio, Presidente, siamo a fine legislatura, siamo tutti grandi

il motivo per cui ho presentato gli ordini del giorno è esattamente figlio delle considerazioni svolte da chi mi ha preceduto - il senatore Palma e il senatore Caliendo - cioè

e quindi per cercare davvero di risolvere un problema e non riproporlo. Il tema relativo al blocco dell'eredità, affrontato in maniera così brillante dai colleghi che mi hanno preceduto, è uno dei paradigmi sui quali si fonda il nostro parere di negatività su questo testo.

di incidere), ma sicuramente testimoniano l'azione dei senatori di Forza Italia a sostegno di un provvedimento sicuramente giusto e importante ma che viene affrontato in maniera sbagliata. Con questi atti di indirizzo provo a tracciare un'idea di come potevano essere visti i cambiamenti che c'era il tempo di fare ma che non si sono voluti fare e che, in questo momento di attesa che ritorni la legge di bilancio, lo spazio dell'Assemblea consente fortunatamente di affrontare. Se lo avessimo fatto per tempo, avremmo potuto dare un buon risultato

molti dei provvedimenti che avete portato in Aula in questi cinque anni, che sono stati abbozzati ma non finiti. Si affrontano i temi ma non si danno le soluzioni, si aprono nuove situazioni che forse in certi casi, sono anche peggiori rispetto a quelle che si volevano affrontare. Spero quindi, per lo meno, nel recepimento dei miei ordini del giorno come testimonianza ed impegno che si poteva fare di più e meglio e quindi auspico il parere favorevole della relatrice e del Governo. *(Applausi

l'ordine del giorno G1.200 del senatore Caliendo sostituirebbe tutta una serie di emendamenti, esclusi quelli all'articolo 5, nel testo

fa, lo definite crimine domestico e intervenite a favore degli orfani; se invece l'assassino è uno *stalker*, un molestatore, una persona che comunque non ha quelle qualifiche, l'orfano non ha nessun tipo di assistenza.

Ma la prova non è sul bambino, che sarebbe oggettiva (i bambini sono rimasti orfani); se c'è un omicidio stradale in cui sono morti il papà e la mamma e rimangono due bambini orfani, io dico: assistiamoli; c'è uno *stalker* che ammazza padre e madre e i figli sono rimasti orfani, assistiamoli. No, non assistiamo quelli, ma assistiamo il bambino che ha ancora il padre o ancora la madre, che rientra in questa categoria e in questa classifica. È, quindi, una legge discriminatoria, assolutamente e ideologicamente discriminatoria.

essere. Quindi boccerete il mio emendamento, che dice che tutti i bambini che rimangono orfani a causa di un omicidio devono essere trattati esattamente in uguale, e farete passare la vostra classifica ideologica, per cui gli orfani hanno diritto a essere assistiti a seconda della qualifica dell'assassino: è un'aberrazione. E, se permettete, una volta bocciato questo emendamento, io di aberrazioni non ne voto, perché poi ci sarà, come sempre, giustamente, un dibattito nel Paese e, quando leggeranno questa norma e capiteranno i primi casi, in cui i bambini orfani non avranno alcuna assistenza, questo vostro manifesto ideologico, come al solito, si rivolgerà contro di voi.

È comune opinione che si voglia tutelare il minore, si vogliano tutelare i figli traumatizzati da qualcosa di importante, negativo, avvenuto in famiglia, in famiglia, nell'ambito domestico. Provo a spiegare, in modo forse più pacato rispetto all'enfasi che ha messo il collega Giovanardi.

in quel caso il figlio non avrebbe le stesse tutele. Quindi, se perde un genitore, per causa dell'altro genitore, rientra in questa fattispecie, se li perde entrambi a causa non di un suo genitore, ma di un ex marito, un ex compagno o una ex compagna, in questo caso è privo di tutela.

Il cerchio non chiude. Noi voteremo a favore, ma auspichiamo che vi sia un minimo di buon senso e che si possa approvare questo emendamento. Presidente, mi sono deciso ad intervenire perché tanto il collega Giovanardi quanto il collega Divina hanno svolto riflessioni che ripropongono un tema centrale anche nella qualità della produzione legislativa che consegniamo al Paese. sui quotidiani qualche riflessione di resipiscenza da parte del Ministro della salute, in relazione alle che lascia aperta la porta a quel dibattito che avevamo promosso finanche in Commissione, ancor prima che in Aula, per correggere storture evidenti, relative all'obiezione. Nitto Palma ha fatto un intervento puntuale e preciso: ci stiamo accontentando del meno peggio, cioè della possibilità di approvare una legge esclusivamente perché c'è la tagliola del tempo e quindi sostanzialmente di approvarla purché sia, nella consapevolezza che stiamo facendo un errore grossolano. grossolano. Mi stupisce ancora di più - me lo permetteranno i colleghi della maggioranza e, in particolare, il Governo e la collega relatrice - una parola di riflessione e di commento rispetto a quanto è stato oggettivamente e obiettivamente osservato come punto di criticità. Ora vorrei chiedere questo: è vero, fra qualche ora finisce questa legislatura; siamo alle prese

un ordine del giorno d'impegno, chiaro, puntuale e preciso. Non mi pare un buon modo di legiferare e comunque, in relazione a ciò, chiedo al collega Giovanardi che autorizzi l'apposizione della mia firma a quest'emendamento, quest'emendamento, che introduce un po' di buonsenso in una legge frettolosa e fatta male. Signor Presidente, vorrei portare un attimo di realtà in questo dibattito che vedo spaziare tra i massimi sistemi, dimenticando che stiamo parlando dell'articolo 1 del disegno

puntualizzare quest'aspetto, anche per ricordare o magari rappresentare all'Assemblea e a tanti colleghi che potrebbero non saperlo che questo beneficio - cioè il fatto che le spese legali nell'assistenza nei giudizi penali o civili da incardinare a tutela di questi soggetti deboli o comunque che si trovino in situazioni di grande debolezza - è in parte solo apparente. Noi non siamo contrari alla disposizione e voteremo favorevolmente all'articolo, però di avere la cortesia di informarvi presso gli operatori del diritto, nella fattispecie gli avvocati, che sono iscritti negli albi del patrocinio a spese dello Stato. Io ne posso parlare, perché ne ho conoscenza diretta e un ricordo molto recente: è uno strazio, perché i pagamenti ai legali sono disposti in misura inferiore alla metà dei parametri, che pure sono acqua fresca; sono corrisposti con notevole ritardo, quando lo sono, e talvolta a distanza di anni

ovviamente, che mi sta ascoltando - è solo apparente e nella sua disfunzione concreta fa sì che molti legali preferiscano non difendere né assistere i soggetti che noi, con

a spese dello Stato, secondo la sua proposta emendativa, debba essere concesso nel caso di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ma, francamente, non capisco l'ipotesi alternativa, che prevede che il beneficio sia concesso

infatti, introducendo in questa nostra conversazione elementi completamente fuori dalla realtà. Un conto, infatti, sono le osservazioni tecniche, che non necessariamente dobbiamo definire errori, ma che possono denunciare il fatto che una legge possa essere scritta meglio e che nel futuro possa anche essere, dopo un corretto

lavori della Commissione sul femminicidio, ma anche chi ha un po' di pratica di questi argomenti, sa bene che gli orfani di femminicidio sono a loro volta vittime di queste storie e che molto spesso la loro vita è da da questa segnata, non solo sul piano economico e delle condizioni di vita, ma anche rispetto all'approccio ai temi della violenza e della tranquillità familiare. Quindi, l'assunto di questa legge è che bisogna intervenire in maniera specifica

e questo elemento della convivenza non c'è, non sarebbe stato il caso di inserirlo in una legge successiva. Questo per dire che le leggi sono sempre perfettibili. Apprezzo molto l'atteggiamento della collega relatrice e dei colleghi che difendono questa legge rispetto al fatto che a fine legislatura

Che poi il gratuito patrocinio sia una questione da discutere, questo lo dice il Buccarella e l'ho vissuto anch'io e so bene che ha ragione. Un'altra cosa che in questo articolo non va bene, a mio modo di vedere, è l'importo: 10.000 euro per il 2017 banalmente oggi possono andare bene, ma per gli anni a venire non vanno bene; però però stabiliscono un principio, quello del gratuito patrocinio, anche in deroga al reddito. Siamo nella condizione di fare un passo in avanti e non possiamo consentirci il lusso di accettare semplificazioni che allontanano dal percorso, introducono introducono elementi di ideologia che alla fine poi a cosa mirano? Apparentemente vogliono eliminare discriminazioni, ma sostanzialmente non riconoscono alla base, sul piano culturale e quindi giuridico, l'opportunità, e io dico la necessità, di tutelare gli orfani di femminicidio.

di monitorare l'effettiva destinazione di risorse finanziarie stanziate per le strutture che si occupano della violenza di genere. Per di più, il testo parlava

beneficio. Noi speriamo che tutte queste risorse siano state usate nel modo migliore possibile, ma il Governo per primo dovrebbe chiedere di monitorare l'uso di queste risorse per quella destinazione e, se non lo volesse fare il Governo, dovrebbe essere il Senato a chiederlo.

fornire dati sul Piano straordinario contro la violenza sessuale di genere approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento, dovrebbe essere una cosa che il Governo fa spontaneamente; dovrebbe cioè essere il Governo a chiederci di farlo, se non fosse

i bambini che rimangono orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato, dal *partner* dell'unione civile o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, ma non è affatto detto che sia il padre del bambino. Anzi: Anzi: il soggetto è l'assassino che ammazza un genitore, ma non c'è scritto da nessuna parte che sia un genitore che ammazza l'altro, perché non si è proprio voluto collegare l'omicidio domestico al fatto che uno sia il padre e l'altro sia la madre. Quindi, può darsi benissimo che una persona risposata, con figli, vada ad ammazzare uno dei due genitori, nel qual caso scatta la norma, anche se non è il padre o la madre, mentre se la stessa cosa la fa il molestatore e ammazza tutti e due i genitori non scatta la norma e non c'è il patrocinio. Ripeto: il soggetto non sono gli orfani.

Dipende dalla qualifica giuridica dell'assassino se gli orfani avranno o non avranno assistenza; questa è una cosa assolutamente inaccettabile e quindi voteremo contro l'articolo 1.

e, per quanto riguarda anche altre fattispecie della legge, tentavano di inserire il concetto della tutela degli orfani dei crimini domestici, anziché la tutela degli adulti in queste variegate situazioni. Ribadisco che la rottura con Forza Italia è stata sulle unioni civili, che era l'unica cosa che da questo disegno di legge non poteva sparire, e non sulla tutela degli orfani, perché è evidente che vogliamo tutelare gli orfani da qualunque parte e da qualsiasi relazione provengano. È prevalsa l'ideologia. Prendo atto che questi emendamenti verranno bocciati e prendo atto che oggi viene fatta un'odiosa discriminazione tra orfano e orfano.

«e della persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza».

si tratti di un fatto importante, perché le modifiche apportate dall'articolo 2 generano una disparità di trattamento evidente sotto il profilo della punibilità

un sequestro conservativo per risarcire dei danni, in tutte le fattispecie che ho citato prima, il pubblico ministero non potrà intervenire in base a questa legge, per assistere gli orfani

valutando la possibilità di estendere anche a minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, orfani di genitori vittime di omicidio, la possibilità di essere tutelati mediante un sequestro conservativo.

Signor Presidente, in questo caso avete sganciato la questione degli orfani dal contesto familiare e dall'attualità della convivenza tra due persone nel caso in cui una sopprima l'altra. Avendo fatto questa operazione e avendo scritto che la legge scatta anche se l'omicida aveva

gli orfani di due genitori piuttosto che correre dietro a questa casistica ideologica che non ha nulla a che fare con gli orfani come soggetti. Quindi anche nell'articolo 4 troviamo un gravissimo errore.

di fare quella correzione, altrimenti i beni dei minori saranno bloccati ed essi non avranno la possibilità di essere aiutati negli studi e nella loro crescita da quei beni. Si può prevedere un invito a valutare

fare una considerazione che dovrebbe tranquillizzare anche il senatore Caliendo. Il rilievo che il testo debba prevedere la sospensione del procedimento di successione è corretto perché, come dice il senatore Caliendo, si possono danneggiare gli altri legittimati. Io ritengo, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 512 del codice civile, senatore Caliendo, sia possibile per l'autorità giudiziaria accedere all'istituto della separazione dei beni della successione. Come orientamento giurisprudenziale, quindi, mi permetto di lasciare agli atti di questa discussione questa nostra volontà che vi sia la sospensione della successione relativamente alla posizione dell'assassino, ma non già degli altri soggetti interessati alla successione. E ben può l'autorità giudiziaria procedere alla separazione dei beni e sospendere la successione relativamente alla quota spettante all'assassino. L'obiettivo è quello di dare, fin da ora, un'interpretazione giurisprudenziale della norma che può essere utile all'operatore.

chiederei, tralasciando l'emendamento 8.4, che almeno si valuti la possibilità di inserire, oltre a misure di sostegno, anche misure agevolative.

caso, che il fine sia chiaro. L'idea è quella di riuscire a predisporre realizzazioni di campagne istituzionali. È un atto informativo che credo chiunque in quest'Aula non possa che approvare. considerando che probabilmente anche in questo caso riceverei un parere negativo, chiedo la trasformazione dell'emendamento 8.5 in un ordine del giorno, per prevedere davvero che vi sia l'impegno a fare delle campagne informative. Non credo sia sia indispensabile una spiegazione delle motivazioni e pertanto confido nell'accoglimento della mia richiesta.

due ordini del giorno diversi, entrambi con la dicitura «a valutare l'opportunità

per quanto riguarda l'affidamento dei minori orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 10, il nostro emendamento è molto chiaro: per chi è rimasto orfano di entrambi i genitori perché sono stati uccisi

sia stata cagionata la morte dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dall'altra parte dell'unione civile (anche se è cessata), dal convivente o da persona legata al genitore stesso (anche in passato) da relazione affettiva. Adesso spiegatemi, anche qui, se non si vuole sfiorare il ridicolo, perché la continuazione dei rapporti affettivi degli orfani deve avvenire solo se i genitori sono stati uccisi da soggetti di questo tipo e che magari da vent'anni non avevano più nessun rapporto con loro; se invece i genitori vengono invece uccisi dallo *stalker*, dal molestatore o da qualsiasi altra persona o in un omicidio stradale, il giudice non deve privilegiare l'affidamento nell'ambito degli affetti familiari. Chiedo se qualcuno mi può spiegare questa cosa. Il problema è che è inspiegabile

che non hanno nulla a che fare con responsabilità avvenute fuori da quel nucleo familiare. Quindi, anche questa mi sembra una misura assolutamente eccentrica, sempre per voler ripetere in tutti gli articoli questa casistica. che questa legge non nasce per gli orfani ma serve solo ad accreditare questa casistica. E gli orfani ne fanno le spese.

quello che noi colpiamo è un bersaglio grosso, quando le battaglie si fanno in difesa dei principi costituzionali, dell'articolo 3 della Costituzione,

non riguarda gli omicidi domestici, in ambito domestico. Non riguarda gli orfani, se non parzialmente. Non riguarda il femminicidio. Se vogliamo allargare a tutti, come è stata allargata la fattispecie, il *partner* uomo di un'unione civile che ammazza un altro uomo rientra in questa legge e, quindi, non è femminicidio; o, viceversa, anche una donna che ammazza il marito. Il problema è che qui si è usciti totalmente dall'ambito familiare, nel momento in cui l'omicidio non avviene più fra il padre e la madre del bambino. Si è voluta rifiutare anche l'idea che chi commette un omicidio nei confronti dei genitori, e quindi lascia i bambini orfani, possa godere di questo provvedimento. Si è usciti dall'articolo 3 della Costituzione, si è usciti dal buon senso ci si è impantanati in una surreale casistica. Che uno sia stato sposato e poi abbia divorziato è facile appurarlo; che uno abbia fatto un'unione civile e poi sia uscito dall'unione, è facile da appurare. Mi sapete dire chi sa appurare se una persona trent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale stabile? Chi è che stabilisce se la relazione sentimentale è stabile o meno? Non

perché l'assassino è un molestatore e non un individuo che trent'anni prima aveva avuto una supposta relazione sentimentale, che non c'è più. Come non c'è più la convivenza;

contributi costruttivi che miglioravano i provvedimenti, non avevo altro da fare che ringraziare l'opposizione per il contributo dato alla qualità amministrativa. Io e la senatrice Cirinnà abbiamo conflitti, ma sicuramente lei non ha

di sconti di pena, di svuota carceri, di pene alternative. Sostanzialmente abbiamo fatto di tutto, tutelato delinquenti e comunque chi aveva commesso i reati e chi era già in prigione lo abbiamo scarcerato. Finalmente, però, a forza di predicare, si va nella direzione da noi sempre auspicata di pensare ogni tanto anche alle vittime e non soltanto a chi commette a chi commette reati. C'è stata abbastanza trasversalità nel valutare le situazioni. Ci siamo augurati che si applicasse il maggior buon senso possibile, e qualcosa di buono

di legge che parlava di inapplicabilità del rito abbreviato per determinati reati, tra cui avevamo inserito anche il femminicidio. Peccato che voi non lo avete voluto trattare in questa legislatura. Avremmo infatti già colmato una parte di questioni che abbiamo anche discusso in questo frangente. Concedendo infatti il rito abbreviato, su chi si macchia di reati, ad esempio di omicidio o uxoricidio, potrebbe arrivare una condanna, derivante dagli

abbiamo voluto definire il femminicidio, anche su stimolo di qualcuno dell'opposizione, perché su argomenti così innovativi dobbiamo avere il coraggio di dare definizioni e di seguirle.

di una situazione che si riverbera sulla serenità dei figli. Parlo con cognizione di causa, per aver vissuto certe situazioni. I figli, quando sono vittime di certe storie, hanno bisogno

Per quanto riguarda invece le altre norme, che pure sono tante e non intendo illustrarle compiutamente, essendo state già illustrate in tanti interventi, i destinatari diretti sono proprio i figli. Mi riferisco - ad esempio - al gratuito patrocinio, su cui sono già intervenuta. Sembra che si intervenga con una norma di tipo economico, ma non è così:

che, molto spesso, è proprio la mancanza di libertà economica che impedisce a tante donne, a tante persone di lasciare l'alveo familiare e di rifarsi una vita, magari perché

non secondo i canoni tradizionali che prevedono la discrezionalità e la mancanza di reddito, ma anche in deroga. Altre norme intervengono a tutela dei minori: parliamo del sequestro conservativo della provvisionale,

qualche giorno fa in audizione, ha potuto fare i conti con dati statistici che ci consegnano una povertà di condizioni dei minori vittime di femminicidi alla quale bisogna dare

vive in una condizione di vita dalla quale difficilmente esce senza alcun sostegno. E sostegno significa servizi, significa assistenza medico-psicologica: tutte cose che che talvolta vengono organizzate a macchia di leopardo in questa nostra strana Nazione in cui in alcune Regioni c'è più sensibilità che in altre. In questo caso, invece, sono previste e disciplinate come servizi da apprezzare sul territorio in maniera gratuita. Certo, quando diciamo in maniera gratuita, sia per il gratuito patrocinio che per l'assistenza medico-psicologica, dobbiamo fare i conti con le somme che sono state messe a disposizione, che sono soltanto simboliche. Noi non abbiamo presentato emendamenti - lo dicevo prima parlando del gratuito patrocinio - perché ci rendiamo conto che dobbiamo approvare oggi un disegno di legge che non è una legge bandiera, dato che introduce principi per noi fondamentali. Ci

non in maniera formale e sostanziale, con un sostegno, ma con un problema in più. Quei bambini, ovviamente, non hanno quel sostegno economico e psicologico che invece la legge deve garantire.

uscire da una famiglia in cui magari è solo il padre o la madre - normalmente, ahimè, il padre - l'elemento che degenera rispetto a un contesto familiare che, per altri versi, è

Il riferimento che è stato fatto, invece, al testamento biologico mi sembra assolutamente improprio. I Ministri della Repubblica giurano sulla Costituzione e sono tenuti a osservare e a rispettare - rispettare - i risultati

un sì a questo provvedimento sul quale abbiamo lavorato e che si basa su principi per i quali ci siamo spesi in tanti momenti di questa legislatura, in tanti ruoli, che ci vedranno, come cittadini e come politici, vigili anche nella fase successiva e futura.

parlamentare e un uomo fondamentalmente onesto intellettualmente e, quindi, una risposta alle sue osservazioni cerco di darla, anche se mi rendo conto che convincerlo è impresa alquanto ardua. Ma a me le imprese ardue non hanno mai spaventato. Il primo punto che vorrei che il senatore Giovanardi considerasse è che vi è una differenza sostanziale - come diceva anche la senatrice Lo Moro nel suo intervento in discussione generale tra la condizione del minore che rimane orfano per effetto di un omicidio consumato dall'altro coniuge o comunque da un soggetto con il quale la mamma ha avuto una relazione

Nel primo caso, invece, il minore si trova a vivere una condizione psicologica completamente diversa, perché ha un legame affettivo con l'assassino e, nel momento in cui viene uccisa la mamma,

al caso in cui il minore non ha alcuna relazione con l'assassino, essendo un soggetto che ha avuto una relazione pregressa

ci ho provato e ci provo, ma credo con scarsissimi risultati. Per quanto riguarda tutti gli altri argomenti del sequestro conservativo, vorrei far notare ai colleghi che pure hanno mosso siffatte questioni che, nel momento in cui c'è la costituzione di parte civile nel processo penale, si realizza un innesto del procedimento civile regolamentato dalle norme del codice di procedura civile nell'ambito del processo penale. Non è esclusa la possibilità dal nostro codice, per la parte civile, di chiedere il sequestro conservativo dei beni del soggetto che si sta processando. Che cosa si è fatto? Si è attribuita al pubblico ministero la stessa facoltà che già già appartiene alla parte offesa, la quale, nel momento in cui si costituisce nel procedimento penale, ben può chiedere il sequestro conservativo e, sussistendone i presupposti, è il giudice penale che, nel rispetto delle regole del processo civile, concede la misura cautelare.

Anche in quel caso è possibile la separazione dei beni della successione per consentire, poi, eventualmente, il congelamento di quella quota di successione spettante all'assassino che, in caso ovviamente di condanna definitiva - sarà ovviamente per indegnità a succedere - viene devoluta agli altri soggetti della successione. Anche in questo caso, le osservazioni si vanificano, perché ben possono il curatore e il giudice della successione procedere alla separazione, ai sensi dell'articolo 512 del codice civile. A questo punto, rimane un testo che vuole in qualche modo esprimere la sensibilità del Parlamento nei confronti di minori che vivono una condizione psicologica drammatica. E, badate, c'è una grande differenza. È stato scientificamente accertato - per esempio - che il minore adottato va alla ricerca dei suoi genitori biologici perché vuole capire e superare quel senso di colpa derivante dal ritenere che è stato abbandonato probabilmente anche per una qualche sua colpa. Anche nel caso del femminicidio, si può verificare questa condizione psicologica nel minore. Il minore - è stato accertato scientificamente - prova la sensazione

lui delle responsabilità e delle colpe. Pensate alla differenza: sensi di colpa in questa direzione

Io penso che con riferimento a questo bambino non vi siano norme della Costituzione che vengono richiamate (articolo 3 e quant'altro), perché le due posizioni soggettive sono completamente differenti.

la corretta distinzione tra le due posizioni e ritenere la norma legittimamente aderente al dettato costituzionale. Per queste ragioni, noi,

Innanzitutto, vorrei fare un'importante riflessione, che tutti hanno già fatto. Si tratta di orfani che sono vittime due volte: la prima, perché si trovano improvvisamente senza punti di riferimento, sia la propria madre, sia il proprio padre; la seconda, perché devono trovare da soli il modo di affrontare una nuova, inimmaginabile e improvvisa situazione e andare avanti con la propria vita, indipendentemente dall'età e dalla possibilità economica. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a licenziare ha l'obiettivo, quindi, di rafforzare e anticipare soprattutto le tutele, rispetto alla condanna definitiva del reo, per i figli rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, a seguito di un crimine domestico, commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, o da un convivente nei confronti dell'altro. Negli ultimi dieci anni, gli orfani dei crimini domestici sono stati circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani hanno perso anche il padre, o perché suicida o perché recluso, e sono stati affidati ai nonni materni, agli zii, o spesso dati in adozione. Negli ultimi trent'anni, si ritiene che siano stati almeno 1.500 gli orfani di femminicidio, di crimini domestici, che non hanno trovato - per così dire - attenzione nelle famiglie parentali, in quanto in difficoltà economiche. La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, ormai strutturale, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sui piani culturale e giudiziario. Al contempo, le istituzioni devono farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime, aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di dare risposte puntuali e celeri,

Come è stato più volte ricordato, si introduce il gratuito patrocinio alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito. Si è intervenuti, inoltre, a equiparare l'aggravante, per l'omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi. E riteniamo questo un elemento qualificante, criticato da alcuni. Riteniamo che debba essere affermata la responsabilità piena degli autori di reato. Non capiamo perché, se esiste un'aggravante per la qualità delle relazioni oggi per gli ascendenti e discendenti, cioè a carico dei genitori o dei figli, questa non debba essere riconosciuta anche nei confronti del coniuge, come se - diciamo in un retaggio culturale - l'uccisione del coniuge venisse ritenuto un omicidio di serie B, quindi meno grave dell'uccisione di un genitore o di un figlio, come se ci fosse una corresponsabilità della vittima dell'omicidio. La legge introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisionale senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, anticipando quindi un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva. Sono state previste anche la sospensione di indegnità a succedere verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, senza aspettare la conclusione del processo. Sono state introdotte nuove norme a sostegno delle vittime e delle famiglie che se ne fanno carico, e in particolare: l'assistenza medico-psicologica gratuita; l'accesso gratuito alle spese sanitarie farmaceutiche; la possibilità di garantire la continuità della relaziona affettiva e quindi, in caso di affidi o adozioni, di privilegiare l'affido e l'adozione verso le famiglie parentali o verso quelle famiglie presso le quali c'è comunque una relazione forte da parte dei ragazzi, che già hanno subito un grave danno e hanno, nella maggior parte dei casi, assistito alla violenza e all'uccisione del proprio genitore. Altre misure significative riguardano la decadenza dell'autore di crimini domestici dall'assegnazione di alloggio pubblico e la possibilità di accedere a una procedura agevolata per il cambio del cognome. Questa norma, che può sembrare banale, ma che in realtà in molti casi consente agli orfani di femminicidio di poter chiudere una pagina veramente dolorosa - se veramente si possa mai dire che possa essere chiusa - e ricostituirsi anche una vita con nuova dignità, con una nuova identità anche attraverso il cambio del cognome. Con la presente proposta di legge ci si pone quindi l'obiettivo di anticipare, a favore dei figli della vittima di omicidio, una serie di tutele che attualmente il nostro ordinamento riconosce solo a seguito di condanna penale in via definitiva e solo a seguito dell'avvio di ulteriori procedimenti in sede civile, con grave penalizzazione degli orfani della vittima, che si vedono riconosciuti pienamente i propri diritti solo a distanza di decenni dal tragico evento che ha cambiato loro radicalmente la vita sia sul piano affettivo che sul piano delle prospettive di vita, anche economica. Si intende inoltre brevemente sottolineare come comunque in questa legislatura siano stati fatti grandi passi in avanti per mettere al centro le vittime nel nostro ordinamento: la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è stato il primo provvedimento approvato nel 2013, il decreto legislativo n. 212 del 2015, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 29 del 2012 in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso norme minime, che assicurano adeguati livelli di tutela e assistenza sia nelle fasi di processo e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. La stessa direttiva prevede inoltre, agli articoli 8 e 9, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, nonché l'assistenza prestata dai servizi appunto di informazione, orientamento e consulenza e accesso ai servizi per le vittime di reati intenzionali violenti. Altri provvedimenti sono legati sempre all'attuazione di direttive europee, tra cui l'indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, a cui noi oggi ci agganciamo anche per sostenere il fondo e le spese di questa proposta di legge. Noi riteniamo che appunto questo provvedimento sia di particolare importanza. È un aggiornamento del quadro normativo che consente una tutela immediata del minore che deve essere tutelato in tutti molteplici aspetti evidenziati nel mio breve intervento. Pertanto, non posso che ribadire il pieno sostegno e il voto favorevole da parte del Gruppo di Alternativa Popolare.

che mi dichiaro soddisfatto, molto contento, del fatto che questo provvedimento arrivi alla fine di questa legislatura

un dovere che oggi lo Stato decide di assumere, impegnandosi, anche con tanti ordini del giorno, per qualificare, monitorare e migliorare l'operatività di una legge necessaria a tutela dei minori vittime delle più intollerabili violenze verso la propria madre e nell'ambito dei rapporti familiari.

Un percorso partito, fatemelo ricordare, dalla Sardegna, fatto di tante tappe: dalla predisposizione del testo del proponente alla Camera, il collega ed amico Roberto Cappelli, al quale ha lavorato sin dall'inizio l'avvocato Anna Maria Busia; un testo diffuso e difeso nel nostro territorio dalle avvocate Margherita Zurru e Loredana Violi, che tanto si sono impegnate con i centri anti violenza in Sardegna e in Italia, alla presentazione in Senato di una analoga proposta a mia firma e al dibattito in Senato sul libro «Carezze di sangue» di Maria Francesca Chiappe, una nostra giornalista impegnata sul quotidiano più diffuso in Sardegna. Il libro racconta la triste vicenda di Dina Dore, vittima di femminicidio, che lascia una figlia, allora neonata,

alla relatrice Cirinnà; tutte le senatrici che hanno svolto in Assemblea un lavoro comune, di discussione e ai fini dell'approvazione: le ringrazio tutte. Ringrazio il Governo, il presidente Grasso, che ha sostenuto l'esigenza di completare l'*iter* legislativo oggi; il Presidente

dimostrandola concretamente ai parenti delle vittime, alcuni dei quali voglio citare a titolo d'esempio: Graziella Dore, sorella di Dina, Mariangela Sedda, sorella di Maria Pina, e Agostino Mele, fratello di Annamaria. Oggi si scrive una bellissima pagina parlamentare, una delle tante bellissime pagine parlamentari che si sono scritte in questa legislatura in termini di diritti e tutele. Questo è stato possibile perché in questa legislatura, in questo tempo, si è deciso finalmente di andare con grande determinazione

sui crimini domestici, ma è un provvedimento contro il femminicidio, contro quella cultura di violenza dell'uomo verso la donna, che passa anche sopra i propri figli, che passa anche sui diritti dei minori. Ringrazio tutti per questo risultato, un regalo bellissimo che credo il Senato abbia voluto rivolgere alla società italiana alla vigilia del Natale. la presente proposta di legge è volta, da un lato, a introdurre misure per tutelare direttamente gli orfani del genitore ucciso per mano del suo *partner* o ex e, dall'altro, a escludere il reo da qualsiasi beneficio successorio o previdenziale che possa derivargli dall'evento mortale che ha causato: obiettivi che sono da noi ampiamente condivisi. In particolare, apprezziamo il fatto

cosa che nel testo originario non era presente e che, anche mediante emendamenti del Movimento 5 Stelle, si è riusciti a inserire durante i lavori alla Camera. Di particolare interesse risulta la norma che prevede la sospensione dell'eredità dell'indagato per l'omicidio del *partner* e l'indegnità a succedere in caso di condanna, anche nell'ipotesi di patteggiamento della pena; indegnità fino a oggi riconosciuta soltanto in sede civile per iniziativa di un altro erede. Condivisibile è anche la norma che introduce la sospensione della pensione di reversibilità dell'indagato per uxoricidio, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, e il riconoscimento di essa agli orfani minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti. Purtroppo - dobbiamo dirlo - l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso, naturalmente. Questo ci lascia in qualche modo non completamente soddisfatti, perché il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con un'educazione volta ad arginare siffatti fenomeni e a tutelare maggiormente tutte quelle donne che invano denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse persone, per mano delle quali verranno poi uccise. Dico questo perché anche se il provvedimento è trasversale - cioè non fa differenza se la vittima di crimini domestici sia uomo o donna - non possiamo non evidenziare che nel maggior numero dei casi vittima del proprio *partner* è proprio la donna. Il Governo all'inizio di questa legislatura, ad agosto del 2013, ha varato un decreto-legge per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quel provvedimento non ha dato i risultati sperati. I dati del Ministero dell'interno sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano 774 casi di omicidio di donne, una media di circa 150 all'anno. Significa che in Italia, ogni due giorni circa, viene uccisa una donna da parte del *partner*. La violenza di genere, purtroppo, provoca vittime anche tra chi resta: un dramma nel dramma. Nel 2014, il 65 per cento dei figli di coppie all'interno delle quali è avvenuta una violenza avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che, dal 2000 ad oggi, gli orfani di femminicidio sono 1.628, di cui 417 solo nel corso degli ultimi tre anni. Tornando al provvedimento in oggetto, riteniamo che, seppur migliorabile in taluni punti, nel complesso esso sia da considerarsi condivisibile ed il testo licenziato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ci è sembrato tutto sommato buono. Certo, avremmo voluto fare di più per tutelare le vittime delle violenze. Avremmo voluto, innanzitutto, mettere una toppa al disastro targato PD nell'approvazione della norma sulle condotte riparatorie, all'interno della riforma del processo penale. Mi riferisco alla norma che prevede che i reati perseguibili a querela soggetta a remissione possano essere estinti tramite un ristoro offerto dall'imputato; ristoro la cui congruità viene valutata dal magistrato ed a cui la vittima non ha alcuna possibilità di opporsi. In questa norma rientravano anche il reato di *stalking* e altri reati contro la persona. Il magistrato può valutare di estinguere il reato quando il reo si attivi per risarcire la vittima, senza che la vittima possa fare alcunché per ottenere che sia fatta giustizia. Tuttavia, abbiamo condiviso l'opportunità di non presentare alcuna proposta emendativa che andasse a riparare i danni causati dalla maggioranza, per non rischiare che il presente provvedimento, costretto a tornare alla Camera a fine legislatura, finisse in un binario morto. Questo perché riteniamo che l'approvazione di un provvedimento che tuteli i figli della vittima di omicidio per mano del *partner* sia, in questo momento, un atto doveroso e di civiltà dal quale non possiamo sottrarci. Comunque, prendiamo atto del fatto che Governo e maggioranza hanno riconosciuto il *vulnus* normativo cui facevo riferimento creatosi con l'entrata in vigore della norma sulle condotte riparatorie e della loro volontà di porvi rimedio, inserendo un apposito emendamento nel decreto fiscale che di recente

sin dall'inizio, quando abbiamo visto questo disegno di legge della Camera dei deputati, il Presidente del mio Gruppo, il senatore Paolo Romani, aveva colto immediatamente un problema di parità di trattamento

terzi non avevano gli stessi diritti. Io non sapevo rispondere quale fosse la ragione di questa disparità di trattamento. Certo, se quel lavoro che abbiamo fatto oggi, quantomeno come raccomandazione per il futuro, fossimo riusciti a farlo in Commissione, forse avremmo potuto varare una legge perfetta, senza alcune sbavature, come abbiamo fatto per i testimoni di giustizia. Mi auguro che, dopo aver approvato il nuovo Regolamento del Senato, vi sia una indicazione di comportamento alle Commissioni su come si deve lavorare

negli stessi termini, perché c'erano alcune cose che gridavano vendetta. Senatrice Puglisi, credo che lei avrà letto

Questo è un modo abbastanza assurdo di lavorare. Dovremmo essere tutti consapevoli che le cose o si fanno con un minimo di calma, attenzione e precisione, altrimenti corriamo questo rischio, perché quell'emendamento incontrava un consenso non formale, ma sostanziale, ed era necessario finanziare quel Fondo. Stiamo votando una legge - e la voteremo - con la consapevolezza degli errori a cui ho fatto riferimento, ma in particolare, per quanto riguarda il bilancio, la copertura del

con cognizione di causa e nell'interesse dei soggetti che si vogliono tutelare. Noi vogliamo tutelare i minori e con questa norma in parte lo facciamo, ma essa necessita di alcune correzioni e mi auguro che la prossima legislatura vi provveda in modo che possono essere tutti tutelati di fronte a reati come l'omicidio volontario, che certamente, da chiunque commesso, determina gravi problemi nella crescita e nella vita

dal dramma dell'uccisione della propria madre per mano del padre, poi suicida nel 30 per cento dei casi o successivamente detenuto. Sono i cosiddetti orfani speciali, 1.600 circa dal 2000 al 2014,

una ricerca importante, in cui, incontrando 123 orfani e le loro famiglie affidatarie, si sono analizzati i loro bisogni a cui noi, con questo provvedimento, intendiamo dare risposta. Dopo tanti anni di silenzio, essi hanno bisogno di attenzioni speciali, di risposte speciali, di tutele speciali e diritti violati da ripristinare. Sono spettatori silenziosi di crimini efferati, nascondono nella mente gli ultimi istanti di vita della donna che ha donato loro la spesso ricordano le sue grida, le richieste di aiuto, il terrore, il silenzio di quando tutto è finito. Le conseguenze di ciò che vivono sono sia di natura fisica che psicologica e psichiatrica, dipendono dall'età dei bambini e da quanta violenza hanno dovuto vivere prima dell'omicidio. cento di queste morti, infatti, arriva dopo molta violenza assistita pregressa. Le reazioni possono essere costruttive o distruttive, cambiano in base al loro carattere. Vivono un trauma nel trauma e il danno che subiscono è esponenziale. Questo provvedimento di civiltà assicura loro assistenza medica psicologica, borse di studio e percorsi di avviamento al lavoro, grazie all'accesso al Fondo, assistenza legale già dalle prima fasi del processo con il gratuito patrocinio. È stabilito inoltre il sequestro conservativo dei beni delle vittime, per rafforzare la tutela degli orfani rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Si mette fine al godimento dell'eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omicidi in famiglia. È una legge perfetta? No, non lo è. Condivido alcune osservazioni del senatore Caliendo, riprese anche dagli interventi in Assemblea del senatore Lo Giudice e della senatrice Lo Moro, ma meglio una legge imperfetta, che nessuna legge, visto che siamo al termine della legislatura. È poi risuonato in quest'Aula un quesito: perché questi orfani meritano una protezione speciale? Perché abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul - questa è la risposta - che riconosce nell'uccisione di una donna in quanto donna una grave violazione dei diritti umani. Essa è giuridicamente vincolante e prevede all'articolo 5 il risarcimento alle vittime, all'articolo 26 protezione

Con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, quindi, non si apporta solo un intervento di ordine sistemico, piuttosto si supera definitivamente l'impostazione del codice Rocco e la sua visione della cittadinanza femminile. Nella prossima legislatura, come chiesto da molti di voi, dovremo estendere questa aggravante anche al coniuge divorziato, alla parte dell'unione civile, ove cessata, per superare questa differenziazione di pena tra coniugi e parti dell'unione civile e divorziati da un lato ed ex conviventi dall'altro. senatore Caliendo, che in realtà il contenuto di quell'emendamento che abbiamo approvato all'unanimità è rimasto intatto. Ne hanno soltanto cambiato il titolo, purtroppo, non so per quale impeto e zelo. e zelo. Con quell'emendamento, che abbiamo approvato all'unanimità, estendiamo a tutti gli orfani di femminicidio, ovvero anche a quelli la cui madre sia stata uccisa in quanto donna da uno stupratore o da uno *stalker*, come purtroppo è accaduto la scorsa estate ad Ester Pasqualoni la dottoressa oncologa di Teramo madre di due figli. Voglio dire anche al senatore Buccarella che quella norma sulla giustizia riparativa e lo *stalking* in realtà l'abbiamo già corretta nel decreto fiscale, quindi siamo già intervenuti riconoscendo un errore che aveva fatto il Parlamento con un intervento del Governo. In questa legislatura abbiamo cercato di affrontare con grande determinazione il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Abbiamo, come dicevo, ratificato subito la Convenzione di Istanbul, subito dopo abbiamo convertito il decreto-legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere che inserisce nel nostro ordinamento misure importanti di protezione e repressione dei reati come il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza a prescindere dalle condizioni di reddito, l'ammonimento e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'arresto in flagranza di reato del maltrattante, l'aggravante per violenza assistita da minori. Per promuovere un vero cambiamento culturale, nella riforma della scuola abbiamo introdotto l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di inserire nei piani triennali dell'offerta formativa azioni di educazione alla parità tra i sessi e di prevenzione alla violenza di genere rivolto non solo a studenti e studentesse ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Recentemente la ministra Fedeli ha emanato le linee guida per l'educazione al rispetto. Nel 2015 è stato presentato dal Governo il Piano nazionale straordinario contro la violenza di genere che istituisce la cabina di regia fra Ministeri, Regioni e istituzioni coinvolte coinvolte nella rete di prevenzione, protezione e repressione dei reati ed un osservatorio cui partecipano anche centri antiviolenza e le forze della società civile. Infine, il 19 aprile il Senato ha istituito la Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, che ho l'onore di presiedere e che a gennaio depositerà, come definito ieri in Commissione, le proprie conclusioni per lasciare indicazioni utili al prossimo Parlamento e al prossimo Governo sulla strada da intraprendere. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare sia la maggioranza che l'opposizione per l'armonia, la serietà e la collaborazione con cui ciascuno sta offrendo il proprio apporto, fatto non scontato con l'avvicinarsi della campagna elettorale e la leale collaborazione anche di tutte le istituzioni al lavoro della nostra inchiesta. Come è emerso dalle indagini ISTAT del 2014, gli autori delle violenze più gravi - violenza fisica o sessuale - sono prevalentemente i *partner* attuali o gli ex *partner* 2.800.000 donne sono state vittime delle loro violenze. Se sono diminuite lievemente le denunce di violenza sessuale (il che non significa che

Mentre il numero di omicidi cala in modo drastico nel nostro Paese e si è ridotto del 39 per cento, la riduzione di vittime di sesso femminile è solo del 14 per cento, come sottolineato dal generale Tullio Del Sette in audizione in Commissione d'inchiesta, questo determina un innalzamento in termini relativi del numero degli omicidi Non solo, ma i dati ci dicono che i delitti sono sempre più efferati. Ma se abbiamo una normativa tra le più avanzate d'Europa, inclusa la legge che oggi stiamo votando, allora perché le donne non denunciano le violenze subite? È questo il grande tema politico che ci dobbiamo porre, sforzandoci sforzandoci di dare le risposte che le donne meritano. Senz'altro occorre offrire percorsi di autonomia abitativa e lavorativa alle donne che vogliamo far uscire dalla violenza domestica, come si è iniziato a fare con il piano straordinario. Occorre la presenza diffusa di centri antiviolenza e case rifugio e la vicinanza delle istituzioni, perché quelle donne con figli possano decidere subito di uscire dalla casa prima che accada il fatto irreparabile. E ancora, come ha ricordato la senatrice Lo Moro nel suo intervento, c'è molto da fare per coordinare il lavoro di magistrati, avvocati e psicologi, assicurando che queste professionalità abbiano un'adeguata formazione

Voglio ricordare qui, perché non fanno parte, purtroppo, di questo provvedimento, anche i 46 bambini uccisi insieme alla madre, 18 uccisi per vendetta verso la ex, fra cui Federico Barakat, ucciso dal padre in un incontro protetto e Andrea Talpis, per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte europea di giustizia per non aver ascoltato le denunce di violenza domestica della madre. madre. È proprio per questo che una delle indicazioni che darà al Parlamento, una raccomandazione che presenterà la Commissione di inchiesta sul femminicidio, è quella di rispettare la Convenzione di Istanbul anche nel caso dell'affido condiviso, che non può essere dato nel nel momento in cui un giudice ha riconosciuto la violenza domestica subita dalla madre e dai suoi figli. Oggi compiamo un passo importante. Sappiamo che forse non è la legge perfetta che avremmo tutti voluto, ma noi la voteremo con grande determinazione perché siamo convinti che quei bambini e quelle bambine, quei ragazzi e quelle ragazze oggi hanno dei diritti in più e quindi

La 12a Commissione, che mi onoro di presiedere, mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, senza modifiche, del disegno di legge in esame. Nel prosieguo dell'esposizione riferirò dunque sul provvedimento quale risultante dopo la lettura della Camera, evidenziando le modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

È evidente che, essendo durato molto l'esame, c'è stato bisogno di un aggiornamento successivo, perché, nel frattempo, si sono fatte

per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché - come aggiunto

e delle menti di uomini e donne, molto importante per quanto riguarda proprio i farmaci. Pensiamo ai *trials* clinici, fatti prevalentemente su una popolazione maschile. Pensiamo, quindi, a farmaci che non sempre hanno lo stesso effetto - anzi, quasi mai - sugli uomini e sulle donne. Ciò dovrebbe essere normale, ma non lo è, tanto è vero che inserire la medicina di genere significa esattamente questo, cioè consentire l'immissione nel mercato di farmaci rispettosi. Faccio solo l'esempio delle malattie cardiovascolari. Di solito si tende a pensare che si tratti di malattie prevalentemente maschili, ma non è più così. Tuttavia, sappiamo che i farmaci sono testati prevalentemente sui maschi. L'osteoporosi viene considerata normalmente una malattia tipicamente femminile. Sappiamo che non è così, eppure i farmaci per l'osteoporosi sono testati fondamentalmente sulle donne. Si tratta, quindi, di una norma - quella sulla medicina di genere - che ristabilisce quella differenza così importante, anche come valore della medicina, dal punto di vista della formazione, in un'ottica *mainstream* (quindi non facoltà specifiche, ma la possibilità di un approccio di genere in tutta la disciplina medica e nella disciplina scientifica). una revisione della disciplina degli ordini e delle professioni sanitarie, che in parte è stata modificata; in particolare, si parla della strutturazione degli ordini professionali e degli ordini sul territorio, delle relazioni tra tra le federazioni e dei codici deontologici. L'articolo 5 inserisce all'interno del sistema sanitario nazionale l'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale),

disciplina integrata, che contempla i due aspetti, sia sociale che sanitario. L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Sappiamo che è un problema, perché molte professioni premono ed era giusto dare un protocollo che consentisse, nel tempo, un percorso lineare per l'eventuale inserimento di professioni all'interno del Servizio sanitario nazionale. che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, altra cosa di straordinario rilievo per il nostro Paese. Voglio solo ricordare che, da una recente ricerca, le persone che si curano con l'osteopatia in Italia sono circa 10 milioni, quindi parliamo di un fenomeno molto ampio. È importante che, accanto all'individuazione della professione, vi sia tutto il normale

nonché, poi, la predisposizione del percorso formativo e delle eventuali equipollenze. Le altre grandi professioni rimangono inalterate. Voglio ricordare che la novità di questo disegno di legge di delega sta

quello dei tecnici di radiologia medica, entro cui saranno collocati gli albi delle professioni che contengono meno professionisti, ossia che sono minori nel senso che sono più piccole, ma non per questo meno importanti. Penso, ad esempio, ai fisioterapisti, ai podologi, agli igienisti dentali, ai logopedisti. Tutte queste professioni potranno avere finalmente un albo

Proseguo velocemente, perché le cose sono davvero tante. L'articolo 11 reca la novella rispetto al Comitato strategico del Sistema nazionale delle linea guida, cosa importante relativamente alla legge sulla responsabilità professionale. L'articolo 12 parla del reato di esercizio abusivo della professione ed è di straordinaria importanza perché l'abusivismo professionale è veramente una delle piaghe che dobbiamo combattere, soprattutto nel campo della sanità. Permettetemi soltanto di citare un articolo prima di concludere, sapendo che ci sono, poi, gli articoli che parlano della dirigenza del Ministero della salute e della disciplina del punteggio massimo dei titoli

per tutti coloro che non chiamerei professionisti, ma personale che in modo scellerato agisce violenza nei confronti delle persone anziane, dei bambini, dei disabili e delle persone più deboli all'interno delle strutture. *(Applausi della penso che questo sia un disegno di legge delega molto importante e mi auguro possa essere condiviso, perché davvero consentirà al massimo di poter lavorare meglio nel Servizio sanitario e di rispondere a più di un milione di professionisti che da dodici anni aspettano di essere riconosciuti nella loro qualità professionale.

e dei consigli, oltre a una modalità di espletare le elezioni all'interno di questi ultimi molto discutibile. Quindi, la possibilità di diventare Ordini e di dare regole più precise comporterà probabilmente una modalità di azione nel tempo migliore di quanto forse sia stata fino a oggi. legge è normato anche l'abusivismo delle professioni sanitarie, che purtroppo ancora oggi permane in tutto il nostro Paese in maniera diffusa, su vari tipi di professioni sanitarie, a danno delle persone che ne usufruiscono e in generale del nostro sistema, perché è comunque un danno sociale.

Dopodiché, mi viene da dire che il disegno di legge, che si dice essere atteso da dieci anni, va a completare la legge n. 43 del 2006, che riguardava, anch'essa, la riorganizzazione delle professione sanitarie, chiudendo in qualche modo un cerchio. Ne sono contenta. Vorrei ringraziare chi, in questi anni, prima di me, si è speso per arrivare a ottenere il riconoscimento degli Ordini, tra cui

Chiaramente, potevamo fare di più, potevamo fare meglio; questo è vero e, lo abbiamo detto anche in Commissione sanità. Devo dire che ritengo il testo che avevamo mandato alla Camera sicuramente migliore di quello che la Camera ci ha rispedito. È chiaro che c'era la necessità di normare la sperimentazione clinica dei medicinali, l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. Mi concentrerò, però, sui due o tre punti

che ne favorisce sia l'equilibrio di genere che il ricambio generazionale nella rappresentanza. È vero che su questo argomento non tutti gli Ordini dei medici sono stati concordi, ma concordi, ma vi sono alcuni punti che a me hanno interessato molto, che sono l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico. Nella mia attività professionale sono stato sempre molto vicino a queste due categorie e devo dire che sono due categorie che sembrano quasi dei fantasmi,

dei notevoli benefici. I motivi, quindi, per cui l'osteopatia deve essere riconosciuta ormai sono abbastanza chiari per tutti. Innanzitutto, per la tutela del professionista osteopata e anche, però, per la tutela del cittadino, che ha bisogno di un diritto alla salute, come dichiarato dalla stessa Costituzione italiana all'articolo 32 e come richiesto dall'Europa. L'osteopatia ha dei modelli di riferimento che la rendono una professione con adeguate evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia. E il costante utilizzo che ne fanno i cittadini per curarsi ne è la conferma. Pertanto, ormai la partita è esclusivamente politica perché documenti ed evidenze di riferimento sono noti a tutti. questo è importante perché con l'osteopatia si curano circa dieci milioni di persone. È vero: sono gli stessi dieci milioni di persone che si rivolgono anche all'agopuntura all'omeopatia. Quindi, io spero che, prima o poi, anche queste figure professionali, che sono sicuramente delle figure professionali di sostegno e di integrazione a livello medico, vengano finalmente riconosciute e accettate anche da questo Parlamento. Ricordiamo che solo nel 1994 viene riconosciuto da parte del Ministero della salute il profilo professionale del fisioterapista. Perché parlo di questo? Perché, fino ad allora, molti fisioterapisti hanno lavorato in una sorta di abusivismo della professione sanitaria. Molti fisioterapisti che ora si pregiano del titolo di professionisti sanitari si sono forse dimenticati che anche la fisioterapia è passata per lo stesso percorso che ora sta impegnando l'osteopatia. La necessità di regolamentare nuove professioni sanitarie, quali l'osteopatia, nasce dall'esigenza di tutelare i cittadini che, in numero sempre maggiore, da venticinque anni ormai la scelgono come sistema di cura. L'osteopatia trova la sua legittimazione in quanto già riconosciuta come professione sanitaria sia dell'Organizzazione mondiale della sanità che dal CEM è approvata nel marzo del 2015 dall'Unione europea in linea e a sostegno del percorso intrapreso dal Ministero della salute, che inquadra l'osteopatia tra le professioni sanitarie con una formazione universitaria. Ho lavorato e sostenuto questa scelta in Commissione perché credo che, in modo illuminato e competente, dobbiamo sostenere le giuste cause che tutelano il cittadino aprono la strada verso una possibile e auspicabile integrazione tra le professioni sanitarie, avendo come fine ultimo la salute del paziente all'interno di un sistema integrato fra ruoli diversi e complementari. legge sono stati approvati in Commissione anche due ordini del giorno da me presentati per il riconoscimento del laureato in scienze motorie tra le professioni sanitarie. Conosciamo tutti il valore degli ordini del giorno, ma credo sia venuto il momento di non ignorare più la figura del dottore in scienze motorie, che, con le sue diverse specializzazioni, è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione della salute nei diversi ambiti, senza nessun riconoscimento professionale da parte dello Stato. Pensiamo quindi non solo all'educazione motoria a scuola (che a mio avviso deve raggiungere i livelli dei sistemi scolastici del Nord Europa), ma anche ai centri *fitness*, alle palestre, alle strutture sanitarie, alle associazioni sportive. Quando si Quando si parla di salute non possiamo affidarci a personale non qualificato e questo è un problema serio, perché, soprattutto nelle prime fasce d'età, l'educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce gravemente sullo sviluppo e sulla salute del bambino e di conseguenza dell'adulto. Inoltre ci viene detto che ogni euro speso in prevenzione tramite una corretta educazione motoria consente di risparmiare oltre quattro euro di spese sanitarie. Nonostante il fatto che i laureati in scienze motorie impiegati sul mercato del lavoro continuano a vantare un tasso di occupazione superiore alla media, uno dei punti più critici è rappresentato dall'elevatissima quota di lavoro sommerso. La percentuale di laureati con contratto a tempo indeterminato è infatti molto bassa. A complicare la situazione c'è poi il problema della condivisione degli spazi con fisioterapisti, una storica guerriglia fatta di invasioni di campo e gelosie professionali: laureati in scienze motorie da una parte, fisioterapisti dall'altra. Anni fa il Parlamento approvò una legge che mise sullo stesso piano le due professioni, ma l'equivalenza scontentò troppi e il Senato la cancellò senza sanare in alcun modo la disparità di trattamento di questi professionisti. Se infatti al dottore di scienze motorie è negata la possibilità di operare come fisioterapista (come ritengo giusto), a quest'ultimo è concesso di operare in ambiti propri del laureato in scienze motorie ed è questo che fanno tanti operatori spesso con competenze tecniche acquisite, ma privi della qualificazione universitaria indispensabile per interventi che riguardano la salute, la prevenzione, i processi educativi e l'equilibrio psicofisico. Detto questo, in parole spicciole e facendo un po' di interpretazione su quanto scritto dal legislatore, il laureato in scienze motorie avrebbe competenze non esclusive e possibilità nelle nelle palestre, nei centri *fitness*, nell'intervento rieducativo, nella preparazione atletica e nell'ambito manageriale. Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che nel decreto legislativo citato non si parla di cosa il laureato in scienze motorie faccia o possa fare, ma in realtà solo delle conoscenze che dovrebbe possedere. È una distinzione che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, poiché vi è differenza tra il possedere delle conoscenze e l'essere l'esecutore unico deputato a mettere in pratica le stesse. Da qui si viene a creare l'equivoco di fondo del laureato in scienze motorie, custode di conoscenze messe poi in atto da chiunque. Pertanto, l'inserimento e la pratica dell'educazione fisica all'interno delle all'interno delle scuole non deve essere più un mero ideale, ma un fatto concreto, vista l'importanza fondamentale che il movimento riveste per l'armonico sviluppo psicocorporeo nell'età evolutiva. Devo dire che ho contribuito a questo percorso, sono contento che il disegno di legge sia arrivato all'esame dell'Assemblea e che venga approvato dalla maggior parte di noi, ma sarei molto contento che anche quest'ordine del giorno si trasformasse in una cosa reale e non solo in parole

mi hanno evidenziato molte considerazioni e segnalazioni, ma una in particolare, quella del signor Antonio, la considero molto interessante e motivata e ve la vorrei leggere: di legge Lorenzin è un'ennesima proposta di legge inutile, anzi dannosa, infatti non rappresenta uno strumento per rinnovare le professioni sanitarie e nemmeno configura in Ordine le dette professioni sanitarie. Continua con il consueto atteggiamento clientelare a proporre contentini per quella o quell'altra *lobby*. Non c'è nessuna attenzione concreta alla tutela della salute pubblica, non si affrontano i veri problemi della sanità italiana. Come al solito il metodo della Lorenzin è coercitivo senza alcun coinvolgimento delle professioni sanitarie. In chiusura di legislatura non è corretto portare avanti norme finalizzate ad agevolare le solite categorie, per non parlare della disgustosa norma dei medici del Ministero della salute (articolo 17) nominati di colpo dirigenti. Articolo che è stato più volte dichiarato incostituzionale e da ultimo dalla 1a Commissione, affari costituzionali, della Camera. La Lorenzin non ricorda che varie trasmissioni televisive (la trasmissione «Report» del 2 dicembre 2013 che parla del famoso emendamento Polverini sonoramente bocciato non è bastata! e testate giornalistiche hanno già denunciato la vergogna di tale iniziativa che altro non è che un ricatto elettorale». Vediamo cosa dice questo articolo 17, che alla prima lettura del Senato era entrato come 13 ed è uscito come 14 e alla Camera è entrato come 14

legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la creazione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri». valutazione non sono al corrente, però è veramente interessante vedere come è stato tradotto l'emendamento Polverini in questo articolo 17 ed è veramente un capolavoro:

Qui sorge la domanda spontanea: come fa a non determinare una maggior spesa se aumentano lo stipendio a 400 dirigenti? Ma vediamo cosa diceva la trasmissione «Report» di cui autore è il giornalista Mottola:

riguardava circa 400 medici, farmacisti, biologi e psicologi che lavoravano al Ministero della salute come dirigenti sanitari e che guadagnavano circa 100.000 euro La Polverini propone, con questo emendamento, che vengano posti sullo stesso livello dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale arrivando a guadagnare fino a 180.000 euro responsabile della funzione pubblica della CGIL, afferma che, dal punto di vista concreto, per la salute dei cittadini, questo intervento non migliora la funzionalità del Ministero della salute e non ci sarà alcun cambiamento per i cittadini. Inoltre, afferma che sarà il prossimo contratto nazionale di lavoro che dovrà pagare il costo di questo emendamento, che quindi è a carico della collettività. Quest'emendamento ha però un percorso assai tormentato e nel settembre 2013, dopo essere stato infilato del decreto per la razionalizzazione, viene giudicato inammissibile. A questo punto l'emendamento viene presentato al Senato, questa volta però dal Partito Democratico. Ma viene di nuovo bocciato, perché giudicato incostituzionale. Dopodiché, ritorna per la terza volta grazie al PdL che lo infila nella legge di stabilità e per la terza volta viene respinto. Interessante anche notare che un comma di questo articolo determinerà un vantaggio per un gruppo ristretto di funzionari, che lo stesso Cosimo Arnone della funzione pubblica della CGIL quantifica in meno di cinque persone: un comma *ad personas*. Finalmente oggi, dopo una gestazione di quattro anni, questo emendamento sarà partorito. Complimenti per la caparbietà! opinabili ce ne sono molte, in questo disegno di legge, anche il fatto, per esempio, che si dà la possibilità a un Albo, su richiesta del suo rappresentante legale, di diventare Ordine. Questo ritengo che dovrebbe essere la maggioranza degli iscritti a richiederlo, perché comporterà una maggiore spesa (spese di segreteria,

che preparano i nostri giovani, i quali vengono illusi e spendono soldi per avere delle scorciatoie per conseguire delle professionalità, che in realtà non hanno. Crediamo quindi che il provvedimento in esame avrebbe dovuto incidere su molte altre criticità, che invece non prende neanche in considerazione.

non smette mai di stupirci, in senso negativo, ovviamente, perché, dopo aver messo in atto una distruzione indiscriminata del nostro territorio, estirpando ulivi, distruggendo campagne dell'intera costa salentina, ora ha iniziato a comprare spazi sulle riviste per farsi pubblicità. L'ultima assurdità, infatti, la vediamo stampata con caratteri bianchi su sfondo verde, sul periodico mensile ufficiale del Sindacato italiano appartenenti polizia

TAP non inquina, perché si limita a trasportare il gas ed è a impatto zero. E ancora, si legge che l'inquinamento dell'aria e le emissioni in Puglia diminuiranno. Hanno pure la sfera magica per prevedere quello sono cose che non esistono, perché questi gasdotti sono bombe ad orologeria, pronte a sterminare non solo l'ecosistema, ma anche le vite umane e lo abbiamo visto anche con l'incidente in Austria. Queste persone hanno letto i giornali di meno di dieci giorni fa, quando si è verificata la pericolosa esplosione all'interno di una stazione di compressione e distribuzione gas? Evidentemente no. Lo sanno che è morta una persona e decine di persone sono rimaste ferite? Evidentemente no. Qui i giornali non li leggono? Lo sanno che quello che è accaduto nel gasdotto austriaco rappresenta un potenziale rischio che potrebbe colpire anche i pugliesi e, più in generale, l'Italia? TAP, diffondendo questi contenuti, comprando spazi pubblicitari ed elargendo corsi di inglese e di cucina, per di più pubblicando su riviste del sindacato di polizia, sta attuando un'opera di disinformazione. Quindi, attenzione! Non cadiamo nella trappola delle bufale di TAP. Se continuano ad avvalersi di pubblicità a pagamento, significa che hanno un disperato bisogno di diffondere delle notizie, delle vere e proprie *fake news*, che gratuitamente non pubblicherebbe nessuno: è evidente! *(Applausi

Oggi, con stupore e anche con contrarietà, ho letto un articolo su «Libero», a firma di Renato Farina, che riporta una serie di insulti, che sono stati rivolti sul *web* nei confronti di Altero

abbiamo letto degli insulti. Quello che avviene in rete e se ne è parlato non ancora abbastanza, è un fenomeno che non ha un colore politico. C'è una parte del saprei neanche se definirlo così), una parte dei cittadini, una parte della popolazione che pensa che questi commenti non lascino alcun segno e invece non è vero. Proprio con il presidente Matteoli abbiamo incardinato un disegno di legge in Commissione 8a a a mia prima firma che ha portato la Commissione ad approfondire un discorso sulla tracciabilità degli autori sulle piattaforme sociali. Abbiamo notato come tale ricerca investigativa sia complessa e difficile. Anche quando il giornalista scrive che sono partite le denunce, non è assolutamente automatico che l'attività investigativa fatta dalle nostre Forze dell'ordine possa portare ad un risultato. Quindi invito tutti ad approfondire questo argomento. Mi piacerebbe che chi riporta commenti

del dottor Giustozzi, del responsabile dei *service provider,* che ci hanno dato elementi importanti. Purtroppo la legislatura è alla sua scadenza e mi dispiace che non siamo riusciti a portare a compimento questo disegno di legge. Io sono sicuro che sia un argomento attuale e che sin dalla prossima legislatura dovrà essere approfondito, perché quello che avviene sul *web,* fatto dai *top player,* è qualcosa di aberrante. è qualcosa di aberrante. Facebook è nato per mettere in comunicazione degli studenti all'interno di un *campus*. Adesso ciò avviene in un altro contesto, ci sono altre regole e soprattutto ci sono altri effetti, quindi

sulle parole non ostili, poi però, quello che avviene sul *web* deve essere regolamentato. Si può mantenere anche il diritto all'anonimato, però persone che